Signor Presidente, onorevoli senatori, a San Pietroburgo, al Vertice G20 del 5 e 6 settembre scorso al quale ho partecipato insieme al ministro Saccomanni, Saccomanni, abbiamo avuto la conferma che, pur tra tanta fatica, l'economia mondiale sta uscendo dalla crisi. Per la prima volta dal 2008, cioè da quando di fatto è nato il G20 in questo formato, non si è discusso infatti di salvataggi,

Per la prima volta il nostro Paese non è stato trattato da sorvegliato speciale, da pericolo per la stabilità dell'Unione europea e dell'intera economia, da recidivo cui assegnare con sufficienza il solito pacchetto di compiti a casa. Siamo arrivati a San Pietroburgo forti del lavoro svolto in questi mesi e in questi anni: un lavoro che è stato foriero di risultati positivi. siamo stati promossi per i risultati raggiunti. Sacrifici e lavoro hanno trovato un ulteriore riconoscimento, e voglio quindi cominciare da questo punto dicendo che questo è stato un grande risultato, un risultato importante, figlio di un lavoro collettivo, figlio del lavoro di questi di questi anni. E posso soltanto permettermi di segnalare con grande forza che questo riconoscimento possiamo rovinarlo in un attimo: basta che buttiamo via la fatica e la stabilità che abbiamo riconquistato faticosamente e ritorniamo facilmente dentro una condizione di grandissima difficoltà. Lo dico in particolare oggi, in un giorno nel quale abbiamo visto e toccato con mano cosa vuol dire che i nostri tassi di interesse, invece di continuare a scendere, come hanno fatto nei mesi scorsi, continuano a soffrire sotto Quello dell'instabilità è un costo pesante per i cittadini, per le imprese, perché è un costo che è pagato in termini di tassi di interesse sul debito. sappiamo tutti, ma lo voglio soltanto ricordare per memoria di ognuno di noi: noi paghiamo ogni anno 85 miliardi di euro non di di debiti ma per mantenere in vita il debito così come esso è; se sbagliamo, quegli 85 diventano 87, 88, 89; se facciamo bene, diventano 81, 80, 79. I tedeschi pagano 20 miliardi meno di noi in termini di peso del debito, i francesi 30 miliardi meno di noi, gli spagnoli addirittura 50 miliardi meno di noi di tassi di interesse sul debito; lo dico perché in quest'Aula, come nell'Aula della Camera ci accapigliamo e discutiamo nelle Commissioni per spostare 10 o 50 milioni da una parte all'altra del bilancio,

ci vuole un attimo soltanto per buttare via tutti i sacrifici che abbiamo fatto e il risultato positivo raggiunto in questi anni. *(Applausi dai all'agenda del G20. La Presidenza russa l'ha fortemente organizzata intorno al tema della crescita, declinando la questione in quattro sessioni di lavoro: l'economia globale, lo sviluppo, il lavoro, il commercio.

Una discussione alla quale ha partecipato, tra l'altro, in rappresentanza delle imprese, una personalità italiana, l'amministratore delegato dell'ENEL, Fulvio Conti. Infine, la Siria, cui è stata dedicata la cena del primo giorno, oltre a numerosi incontri bilaterali. Parto dai *dossier* economici: durante il Vertice sono emerse tutte le differenze tra Paesi emergenti e industrializzati; differenze di posizioni e di prospettiva, che restano profonde. Penso, ad esempio, all'apertura delle frontiere commerciali, agli *spillover* negativi delle politiche monetarie. A fronte di queste divergenze, al G20 si sono però ottenuti sicuramente risultati concreti. È vero, le negoziazioni sono sempre più complicate. Quando però conducono ad un accordo, questo è decisivo e dirimente. Basti pensare ai passi avanti che sono stati fatti sul fronte fiscale (insisto su questo punto): un traguardo

di Cannes) i temi chiave erano invece l'instabilità finanziaria, i salvataggi, le emergenze. Il Piano d'azione del G20 di San Pietroburgo

molto importante. Occorre uscire da quella contrapposizione sterile tra austerità e sviluppo e crescita. Occorre ribadire, ancora una volta, che il rigore fine a sé stesso non basta, se non ci sono accanto politiche per la crescita. Dal G20 tutti i Paesi sono usciti con impegni di politica economica. Per l'Italia essi coincidono in pieno con l'agenda che in questo Parlamento abbiamo insieme definito: l'impegno a dare liquidità alle piccole e medie imprese, pagando rapidamente i debiti della pubblica amministrazione, in linea con quanto il Governo Monti ha deciso qualche mese fa; l'impegno a favorire l'ingresso nel mercato obbligazionario anche delle piccole e medie imprese, che devono essere e rimanere ancora di più al centro della nostra attenzione, con l'estensione dei fondi di garanzia, gli incentivi con gli investimenti di capitale. Ci siamo poi impegnati a lanciare il programma di attrazione degli investimenti che chiamiamo «Destinazione Italia» entro l'autunno, per renderlo operativo al più presto. Ci siamo impegnati a continuare la semplificazione ed il miglioramento della giustizia, in particolare amministrativa e civile, vitali per ridurre i costi di transazione per le imprese. La seconda priorità era il lavoro, soprattutto quello giovanile: un impegno molto forte, a partire dal Consiglio europeo di giugno giugno e dal G8 di luglio. Il G20 ha lanciato un chiaro messaggio, chiedendo a tutti gli Stati di adottare misure per la crescita accompagnate da politiche attive per il lavoro. A questo proposito, ricordo un fatto molto importante: il vertice del G20 per la prima volta ha applicato un metodo

Il vertice che ospitammo a Roma il 14 giugno tra Francia, Italia, Spagna e Germania è stato un vertice tra Ministri delle finanze e del lavoro insieme, un formato che a livello internazionale non si era fino ad ora sviluppato. Insisto tanto su questo punto,

il cuore di tutto è un complesso di politiche economiche in cui i Ministri del lavoro giocano un ruolo fondamentale, perché sono quelli che più di tutti hanno, hanno, alla fine, il contatto con la gente, i lavoratori, le persone che hanno bisogno del rapporto con il *welfare*. Cito questo punto perché l'ho considerato un passo avanti molto importante delle istituzioni internazionali, che guardano devono guardare sempre di più ai temi non soltanto nella centralità degli aspetti finanziari. È un errore immaginare che il cuore di tutto siano le decisioni finanziarie: il cuore di tutto deve essere la somma cercare di mettere insieme i vari aspetti. Sono quindi particolarmente contento che la scelta che abbiamo lanciato qui da Roma sia diventata e stia diventando sempre di più, con il G20, il metodo di lavoro più normale.

alla legge di stabilità e ai prossimi progetti di politica economica. Tagliare il costo del lavoro è il cuore di tutte le politiche per la crescita rispetto al tema del cuneo fiscale. la rapida introduzione della *Youth* *Guarantee*, la riforma dei centri pubblici per l'impiego. Credo che queste siano questioni di grandissima importanza e centralità su cui La terza priorità italiana era la regolazione dello *shadow banking*, di tutto ciò che è finanza ombra ed è fuori dalla regolazione che fino ad oggi invece le istituzioni internazionali sono riuscite a creare. La dichiarazione finale include una tabella di marcia serrata da portare avanti, insieme al Financial Stability Board, entro il 2015. È la prima volta che questo accade, e lo considero un altro passo importante, perché la finanza non sia senza regole, Il quarto obiettivo riguardava la lotta all'evasione fiscale. abbiamo spinto perché entro il 2015 tutti i Paesi del G20 siano obbligati a procedere con il sistema dello scambio automatico delle informazioni, come nuovo standard globale per la lotta all'evasione. È una rivoluzione.

a lottare contro i paradisi fiscali; una lotta che è per noi oggi la grandissima priorità. Lì si vanno a ritrovare le risorse, quelle risorse di capitali italiani su cui non si pagano le tasse in Italia

Sappiamo tutti che su questo tema non ci sono logiche nazionali che contano: o c'è un grande accordo globale ed internazionale oppure i risultati non si riescono a raggiungere. Il quinto obiettivo, sempre sul tema tasse, era quello che toccava era quello che toccava la lotta all'elusione fiscale. Il G20 ha accolto ed approvato un piano molto importante, e lo voglio qui sottolineare perché, come penso sia chiaro a tutti, su questi temi l'attenzione della pubblica opinione, che era ovviamente tutta concentrata sulla Siria, è stata un po' più lasca.

shifting*) ossia tutte quelle norme che consentono alle multinazionali di eludere i meccanismi fiscali tra Paese e Paese, finendo per non pagare le tasse dovute,

l'accordo globale contro la corruzione a livello internazionale. Abbiamo fortemente spinto sull'impegno di tutti i Paesi ad adottare le convenzioni ONU

le condizioni peggiori per la crescita. E un Paese come l'Italia, ad economia aperta per definizione, con il protezionismo finisce per perdere più di tutti gli altri. L'accordo che è stato individuato, di posporre fino al 2016, quindi più di quanto nei testi iniziali era indicato, il blocco di nuove forme di protezionismo lo considero molto, molto importante. Riassumendo, obiettivi centrati ma ancora tanto lavoro da fare. Sul piano strettamente politico il G20 ha costituito un'occasione di dialogo con i Paesi emergenti: penso al Brasile, alla Cina, all'India, al Sudafrica, come pure ad alcuni Paesi definiti Paesi definiti come «i prossimi 11», tra i quali la Corea del Sud, l'Indonesia, il Messico, la Turchia. Da San Pietroburgo è giunta l'opportunità di rafforzare un percorso comune rivolto alla crescita e a un maggiore scambio politico e commerciale. In questa chiave vanno letti gli incontri bilaterali che abbiamo avuto Corea del Sud, Messico, Russia, Cina, Giappone e Singapore. A tutti abbiamo illustrato il cosiddetto piano Destinazione Italia, nella nostra volontà di metterlo a punto - ovviamente non è ancora pronto - e a tutti abbiamo ricordato la grande opportunità di visibilità e interazione offerta da Expo Milano 2015 che anche in quella sede è stata vista - lo è a maggior ragione per noi - come una grandissima e straordinaria opportunità per raccontare il meglio dell'Italia dentro uno

il G20 si è concentrato ovviamente sulla questione della Siria. Su questo tema voglio sviluppare la parte più consistente della mia riflessione insieme a voi. È possibile percorrere la strada della pace? Possiamo uscire da questa spirale di dolore e morte? Solo qualche giorno fa, Papa Francesco ha sollevato dal sagrato della Basilica vaticana questi interrogativi, interrogativi, che sono echeggiati con forza straordinaria e vibrante nella piazza reale di Roma e nella piazza virtuale della comunità internazionale; interrogativi che colpiscono il mondo e ciascuno di noi e impongono risposte all'altezza del dramma smisurato che essi evocano. Su questa spirale di dolore e di morte in Siria, sulle immagini spaventose diffuse dai circuiti internazionali, sulla contabilità incerta e drammatica delle vittime, sui milioni di disperati che giorno dopo giorno transitano oltre i confini di quel Paese, il nostro Governo ha mantenuto e intende mantenere un raccordo trasparente e sistematico con questo Parlamento. Già nelle comunicazioni del 27 agosto presso le Commissioni affari esteri di Camera e Senato il ministro Bonino ha messo in evidenza i capisaldi della nostra posizione. Oggi voglio qui confermare quell'impostazione, aggiornandola naturalmente alla luce di quanto successo. Prima di tutto c'è una condanna netta ed inequivocabile ribadita in ogni consesso nazionale e internazionale, formale e informale, informale, nei confronti dell'utilizzo delle armi chimiche, come quello avvenuto nei dintorni dei quartieri orientali di Damasco lo scorso 21 agosto la censura per un atto che si configura, senza alcun dubbio, come un crimine contro l'umanità che, in quanto tale, esige una sanzione dura, pronta e adeguata da parte della comunità internazionale. È questa, del resto, la posizione dei nostri alleati statunitensi, ai quali ribadiamo la nostra vicinanza e amicizia, particolarmente oggi, 11 settembre, giorno che evoca un dramma che non deve mai più ripetersi. L'uso delle armi chimiche, dicevo, non può diventare un precedente ed è il confine invalicabile; è la negazione stessa del nostro percepirci essere umani in relazione gli uni con gli altri. Per questo, la comunità internazionale deve assumere in pieno le responsabilità che le sono proprie. Per questo, occorre adottare subito misure di deterrenza in grado di prevenire in Siria, nell'intera regione e dovunque il ricorso a questi micidiali strumenti di morte e paura. Questi strumenti, lo ricordo, sono stati banditi dalla coscienza dei popoli, oltre che dal diritto, oltre novant'anni fa. Il secondo pilastro della nostra posizione, ribadita anche a San Pietroburgo, è la centralità del ruolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite quale supremo garante della pace e della sicurezza internazionale. Questa funzione non può né deve essere scalfita. Sono convinto che per il Consiglio di sicurezza dell'ONU esiste ancora lo spazio - angusto ma percorribile - per adottare misure urgenti e incisive capaci di assicurare la messa in sicurezza delle armi chimiche in Siria e di prevenirne l'uso. Dobbiamo appunto percorrerlo, quello spazio. Il nostro Governo sta lavorando, in ogni sede per incoraggiare queste dinamiche sul piano diplomatico, in primo luogo perché crediamo che un'azione militare al di fuori del quadro di legittimità assicurato dalle Nazioni Unite finirà per ingenerare reazioni e controreazioni imprevedibili e pericolose. Per questo abbiamo deciso e comunicato ai nostri alleati che l'Italia non parteciperà ad interventi militari in assenza di un preventivo mandato delle Nazioni Unite. terzo punto è l'impegno per la costruzione di una posizione comune tra i Paesi dell'Unione europea. Ogni crisi internazionale è una sfida per la pace della regione e dei Paesi interessati. Oggi, però, più che mai è anche una sfida per l'Europa, per il futuro dell'Unione europea, in un mondo in straordinaria e complessa trasformazione, una sfida per la nostra politica estera e di sicurezza comune e per la credibilità stessa del progetto comunitario. Ogni Governo europeo ha la propria agenda e i propri condizionamenti esterni: lo sappiamo. Tuttavia, è cruciale che, a dispetto di queste differenze, tutti sappiamo trovare un codice in comune per parlare con una voce sola: la voce dell'Europa, la voce dell'Europa unita. Se non lo facciamo, la pena è certa e senza appello: la condanna all'irrilevanza, una pena altissima che non possiamo e non vogliamo permetterci. È una pena che l'Italia sta cercando e cercherà sempre di sventare, contrastando ogni tentazione di rinazionalizzare le politiche estere, da qualunque parte essa si manifesti. A questi punti, il Ministro degli affari esteri, il Ministro della difesa, il sottoscritto e il Governo tutto si sono attenuti con coerenza, anche nei più recenti sviluppi della vicenda siriana, e li abbiamo promossi in tutti i fori in cui si è articolata la consultazione diplomatica multilaterale. Proprio in funzione di questa impostazione, e in coerenza con quanto affermato finora, va letta quindi l'adesione dell'Italia al documento sottoscritto a margine della riunione del G20 di San Pietroburgo venerdì scorso, sottoscritto da 11 Paesi in quella sede e poi da altri successivamente (Germania in testa). È un documento che quindi è stato sottoscritto da tutti i Paesi europei

che impegna i firmatari europei a lavorare per conseguire una posizione comune europea. Proprio questo riferimento ha aperto la strada al consenso

È una posizione, lo confermo, che si pone in coerenza con la Dichiarazione di San Pietroburgo: anch'essa, infatti, avverte che la comunità internazionale non può restare inerte dinanzi alla barbarie delle armi chimiche ed invoca una chiara e forte risposta. Questi crimini sono inaccettabili e non possono godere di impunità. Fin qui le dichiarazioni di intenti, i comunicati, le parole. Ora dobbiamo operare per trasformare in fatti ciò che dichiariamo. Dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi affinché il Consiglio di sicurezza abbia davvero l'opportunità di adottare misure incisive e di centrare tutti questi obiettivi di deterrenza. Lo spazio per una soluzione alternativa esiste ancora. Negli ultimi due giorni questa opportunità è stata finalmente qualificata da qualche segnale incoraggiante: mi riferisco in particolare alla proposta russa di porre l'arsenale chimico siriano sotto controllo internazionale. L'iniziativa di Mosca e la immediata disponibilità americana, del presidente Obama, a esaminarla lanciano due messaggi. Il primo sul metodo: una soluzione politica resta possibile, come noi abbiamo detto fin dall'inizio. Il secondo sulla sostanza: pur senza condonare le responsabilità per il passato (che gli appropriati organismi internazionali dovranno accertare e comunque sanzionare), la priorità ora è una: evitare che l'uso criminale delle armi chimiche si ripeta. A questi messaggi

di dare seguito alla proposta attraverso meccanismi stringenti di attuazione e di verifica. Attuazione e verifica. Dalle parole ai fatti, Onorevoli senatori, non facciamoci però illusioni. Ho speranza, ma non facciamoci illusioni. La strada diplomatica resta in salita. Per conquistare consistenza è necessario che questa opzione sia corredata di garanzie e di verifiche. Si tratta comunque di una pista, una strada da battere con determinazione e buona volontà. Una strada che rispecchia gli auspici che l'Italia da giorni formula: essendo ormai accertato l'uso delle armi chimiche in Siria, la prima urgenza è uno sforzo della comunità internazionale per sanzionarlo e prevenirne la reiterazione. per New York, insieme al ministro Bonino, per la sessione inaugurale dell'Assemblea delle Nazioni Unite. Lì rilanceremo la scelta italiana a favore della centralità dell'ONU, e sarà l'occasione per contribuire a ulteriori passi avanti nel percorso di pace intrapreso. Dalla questione delle armi chimiche vorrei ora, insieme a voi, allargare lo sguardo su due aspetti più generali che interrogano con analoga urgenza la nostra responsabilità e la nostra stessa coscienza. In primo luogo, le prospettive del conflitto in Siria, al di là della vicenda delle armi chimiche. Siamo e restiamo convinti che nessuna delle parti in conflitto sia in grado di prevalere sul piano militare, né sarebbe in grado di stabilizzare efficacemente il Paese attraverso vittorie sul campo. Una soluzione politica, negoziata, rimane l'unica opzione praticabile per una stabilizzazione duratura della Siria e della regione. Per fare questo, dobbiamo continuare a sostenere la convocazione della Conferenza di Ginevra 2; urgente, indispensabile. Alcuni fattori hanno sinora ritardato l'avvio del processo negoziale, non escluse le incomprensioni tra gli stessi promotori dell'iniziativa. Peraltro, oltre a rivelare i tratti più atroci di una guerra civile, il dramma siriano assume sempre di più i connotati di una guerra per procura, dunque è ora necessario che tutti gli attori che svolgono un ruolo in questa crisi accettino di disinnescare i combattimenti sul territorio. Chiudo su questo punto - e vengo al secondo - condividendo con voi alcune riflessioni sulla risposta cui ci chiama la drammatica emergenza umanitaria. A San Pietroburgo con alcuni Paesi alleati (tra cui il Regno Unito, la Francia, il Canada e il Giappone) abbiamo stabilito di aumentare da subito le risorse per l'emergenza umanitaria, peri profughi, dato che, ad oggi, le agenzie dell'ONU hanno a disposizione fondi pari a meno della metà di quanti ne sarebbero necessari. Insieme abbiamo deciso di intervenire sul piano sanitario a sostegno delle vittime degli agenti chimici; insieme abbiamo valutato la modalità per rimuovere gli ostacoli all'instradamento dell'assistenza umanitaria nel Paese. Sono tre scelte importantissime. Mi soffermo sulla prima, confermandovi che li abbiamo deciso un forte incremento dei contributi al Piano di risposta umanitaria delle Nazioni Unite. Il Governo italiano ha annunciato a San Pietroburgo lo stanziamento di 50 milioni di dollari come ulteriore nostro contributo alla gestione dell'emergenza. Ieri stesso ho parlato sulle modalità di utilizzo di questi 50 milioni di dollari che il Governo italiano proporrà al proporrà al Parlamento di destinare ai profughi e alla gestione dell'emergenza lì, per evitare ovviamente che tutto questo si traduca in un dramma globale ancora più clamoroso, con il direttore esecutivo del *World food programme*, Ertharin Cousin, ribadendo il nostro pieno sostegno al lavoro che le agenzie umanitarie dell'ONU stanno portando avanti nella regione. Dobbiamo alleviare le sofferenze in Siria e degli Stati vicini, sui cui confini si sono già accalcati 2 milioni di profughi. 2 milioni di profughi. Ripeto la cifra perché è impressionante: 2 milioni di profughi. È un intervento essenziale per ragioni umanitarie e per evitare il collasso dell'economia e della società di Paesi la cui stabilità è preziosa per la sicurezza regionale e mondiale. Penso alla Giordania; ma penso anche al Libano, dove opera - e in modo meravigliosamente efficace - un avamposto d'Italia, quel contingente UNIFIL che ci rende, in definitiva, un Paese confinante con la crisi siriana. Onorevoli senatori, due giorni fa a Palazzo Chigi ho avuto il privilegio di ricevere, insieme al vice presidente Alfano e al ministro Bonino, Domenico Quirico, un uomo finalmente libero...

un uomo finalmente libero... *(Applausi)* ...strappato da una terra che invece, purtroppo, continua a nascondere un altro grande italiano, padre Dall'Oglio. Negli occhi di Quirico ho letto la sofferenza di un dramma, che certo è stato individuale, ma che riguarda e investe noi e il nostro stesso ruolo. Dai suoi racconti, dalle sue parole affiora forte, infatti, tutta la complessità del tempo in cui viviamo; una complessità straordinaria, in questo caso tragica, cui abbiamo la responsabilità e il dovere di corrispondere con scelte faticose e coraggiose: scelte all'altezza delle istituzioni che abbiamo l'onore di servire e delle aspettative dei nostri cittadini,

Signor Presidente del Senato, signor Presidente del Consiglio, dividerò in due parti il mio breve intervento, seguendo la traccia dell'informativa del presidente Letta: le prime riflessioni sono sulla dichiarazione finale del Vertice di San Pietroburgo per la crescita e l'occupazione,

poiché tutti noi abbiamo conoscenza della questione e dei termini in cui essa si presenta al Parlamento, ma vorrei riassumere il tutto con una frase: è molto difficile rialzarsi, ma è molto facile compromettere i risultati in un solo momento. Signor Presidente del Consiglio, noi sappiamo che se lei si è presentato a San Pietroburgo con le carte in regola, questo è stato prima di tutto grazie al sacrificio degli italiani e poi allo strumento con cui questi sacrifici si sono realizzati: sono state le azioni conseguenti, coerenti e dolorose, che il governo Monti prima e il governo che ella presiede oggi, coerentemente hanno messo in atto per il risanamento del bilancio pubblico e per il rilancio del nostro Paese. Tutto quello che dovesse intervenire oggi a bloccare questo lavoro, rendendo vani i sacrifici degli italiani, si configurerebbe come un atto di pura irresponsabilità politica. franchezza, guardando in faccia i colleghi degli altri Gruppi politici, ci rendiamo conto che la situazione è delicata per tante ragioni, ragioni, che coinvolgono personalità politiche importanti e fondamentali per alcune aree in particolare; ma noi riteniamo che queste incomprensioni debbano essere superate facendo leva sul rispetto delle regole dello Stato di diritto, sul rispetto che sempre si deve nutrire per i membri del Parlamento, in particolare - per chi tali li ritiene - per gli avversari politici, e che possa responsabilmente compromettere l'esito di questo Governo. Lo sforzo che gli italiani stanno facendo suo tramite non può essere interrotto e, soprattutto, non può essere vanificato. Voglio dire anche un'altra cosa rivolgendomi al ministro Saccomanni. Non mi è piaciuto lo spettacolo estivo di un Ministro che viene tirato per la giacca dagli uni e dagli altri rendendogli ancora più complicato il lavoro che, responsabilmente e con spirito di servizio, sta facendo per il nostro Paese. Voglio esprimere a lei, signor Ministro, la solidarietà mia e del mio Gruppo. Il Governo Letta non è il secondo tempo della nostra campagna elettorale: è un Governo di compromesso politico, perché così è inevitabilmente. Ci sono punti che stanno più a cuore al centrodestra e punti che stanno più a cuore ad altre parti politiche, ma dobbiamo dare a chi ci governa il compito di fare una sintesi, perché se su ogni questione siamo all'ultima spiaggia voi capite che diventa impossibile per chiunque governare, e credo che nessuno, purtroppo, abbia la bacchetta magica. Questo è quasi tutto. Dopodiché siamo d'accordo sul coinvolgimento delle parti sociali, sul fatto che bisogna bisogna abbinare rigore e crescita, sulla necessità che la lotta all'evasione fiscale e alle elusioni venga posta in essere a livello planetario perché

siamo fortemente convinti che bisogna fare uno sforzo per abbassare le tasse sul lavoro. Sul tema del cuneo fiscale l'Italia si è impegnata. Sono importantissime sia che il blocco dell'aumento dell'IVA, ma oggi c'è la necessità di dare un drastico segnale sul tema del cuneo fiscale e delle tasse sul lavoro. Quanto al secondo punto, cioè la Siria, vorrei essere non diplomatico, ma - se è possibile - abbastanza brutale. La posizione italiana è ineccepibile ed è frutto della convergenza tra il Parlamento e il Governo. testimoniare in sede di G20 e in sede di ONU e di Europa una posizione coerente e lineare è stato perché il 27 agosto, nelle Commissioni congiunte affari esteri di Camera e Senato c'è stata una convergenza di tutte le parti politiche. Non ci sono state divisioni tra maggioranza e opposizione, non dico tra destra e sinistra, ma - ripeto - tra maggioranza e opposizione. Non ci sono state diversità. Noi riteniamo che sia un errore politico di primaria grandezza un'azione militare verso la Siria. E voglio essere brutale: qui non c'è uno Stato combattuto da democratici e liberali che vogliono sostituire al despota qualcosa di migliore; qui c'è uno Stato terroristico combattuto da bande terroristiche. Questo è testimoniato in modo straordinario proprio da Domenico Quirico nel suo *reportage* che ha fatto ieri per «La Stampa». Se si fosse intervenuti con preveggenza un anno e mezzo fa si sarebbero evitati i profughi, i morti, ma soprattutto si sarebbe potuta modellare l'opposizione siriana incanalandola secondo binari costruttivi. Questo non si è fatto perché c'è stata un'incertezza, un'inadeguatezza, un'incapacità di visione. Oggi intervenire dopo che tanti crimini sono stati perpetrati, di tutte le nature e di tutte le modalità, con armi chimiche, ma non solo, dal regime e non solo da questo (anche dalle bande terroristiche che al regime si contrappongono) significa andare a incendiare irresponsabilmente ancora di più un Paese.

un coinvolgimento dell'ONU, non ci può essere una nostra presenza in alcuna azione. Ma cosa vuol dire questo? Traduciamolo in parole povere: vuol dire che, se la Russia e gli Stati Uniti non si mettono d'accordo, e cioè l'ONU non si pronuncia, diventa irresponsabile un'azione unilaterale. Essa, tra parentesi, scatenerebbe una sorta di guerra strisciante tra Russia e Stati Uniti sulla vicenda del Medio Oriente, e noi abbiamo bisogno della Russia: abbiamo bisogno della Russia per la Siria, abbiamo bisogno della Russia per l'Iran, abbiamo bisogno della Russia per governare un'area che è di instabilità, perché le primavere primavere arabe ci hanno consegnato una situazione in cui si è dispersa la statualità dei singoli Stati a cui noi eravamo abituati a rapportarci. Questo è capitato in Libia, e diciamo la verità: le riluttanze di Berlusconi erano giuste, allora, e probabilmente non sono state percepite. alla fine oggi che cosa abbiamo? Abbiamo un'instabilità ingovernabile a qualche chilometro dalle nostre coste. Vorrei far notare ai colleghi, poiché io amo il Parlamento e il parlamentarismo,

Parliamo di riforme costituzionali: in un sistema presidenziale per eccellenza il Presidente, capo delle Forze armate, deve parlare con l'ultimo parlamentare. Ma questa non è una debolezza: è la ricchezza della democrazia e del Parlamento di cui noi tante volte non riusciamo ancora in qualche modo in qualche modo ad essere consapevoli. Eppure, questo è il ruolo del Parlamento.

Nella recente riunione del G20 si è discusso della crisi siriana che dura da più di due anni. Sono emerse diverse posizioni fra i venti Paesi e si sono palesate ancora una volta le divisioni esistenti fra le Nazioni europee. Non c'è da essere orgogliosi, per usare un eufemismo, di far parte di un fronte di Paesi europei così frammentato e diviso: la Francia interventista, il Regno Unito frenato dal voto parlamentare, la Germania semplice spettatore e l'Italia in attesa delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, confidando di fatto nel veto di Russia e Cina. Questo deludente risultato non nasce però improvvisamente a San Pietroburgo. È figlio di una incapacità di iniziative positive e propositive su questo conflitto. Mi riferisco alle iniziative diplomatiche che non hanno visto e non vedono tutt'ora protagonisti gli Stati membri dell'Unione europea e in particolare non vedono parte attiva l'Italia, la quale invece, per la sua collocazione geografica, ha forse i maggiori interessi in una soluzione pacifica del conflitto. Abbiamo assistito lo scorso maggio, durante il vertice dei Ministri degli affari esteri, a sconcertanti decisioni pilatesche: prima fra tutte quella di lasciare libertà agli Stati membri relativamente alla vendita di armi dal 1° agosto. Ma poi gli stessi Ministri si sono ritrovati ad agosto a lamentare l'*escalation* militare e il terribile e disumano utilizzo di armi chimiche avvenuto il 21 agosto. Sembrano proprio lacrime di coccodrillo! Le chiedo pertanto fortemente, presidente Letta, di sollecitare un'azione diplomatica più forte e incisiva da parte dell'Unione europea, di cui siamo membri fondatori. Ma le chiedo anche e soprattutto che sia l'azione diplomatica italiana ad essere più forte e incisiva. Non aiutano purtroppo, però, le divergenti posizioni fra lei, Primo Ministro, firmatario della nota degli 11 del G20, che indica nel regime siriano di Assad l'unico responsabile delle armi chimiche, e la Ministra degli affari esteri, che invece resta in attesa del *report* degli ispettori ONU, cui mandato peraltro non prevede l'individuazione dell'autore dell'attacco, ma solo dell'avvenuto attacco. Siamo tutti concordi nel ritenere la via negoziale e del confronto fra le parti coinvolte nel conflitto l'unica possibile Un fronte ampio sostiene questo, un fronte che comprende dal segretario generale della NATO Rasmussen, espressosi in tal senso la settimana scorsa a Vilnius nella Conferenza interparlamentare sulla sicurezza europea, fino a Papa Francesco, le cui iniziative per la pace sono a tutti note. Le azioni militari prospettate anche questa notte dal presidente Obama rischiano invece di compromettere la via negoziale per la risoluzione del conflitto. L'Italia si deve tener fuori dalle azioni militari e, al contrario, adoperarsi per riattivare i canali diplomatici finalizzati alla realizzazione della sospirata Conferenza Conferenza di pace di Ginevra 2; questo nonostante le oggettive difficoltà che ci possano essere. La ministra Bonino, nelle varie occasioni in cui è venuta a riferire in Parlamento, ha dimostrato di avere chiara la pur complessa situazione siriana. Forti anche di questo, chiediamo a lei presidente Letta e al suo Governo più coraggio nell'intraprendere azioni diplomatiche. Ritengo che non manchino all'Italia le possibilità e le capacità in tal senso. L'inazione rischia di diventare complicità. L'Italia deve rafforzare la sua scelta per la via diplomatica con passi e azioni concrete, altrimenti rischia di essere vuota retorica. L'Europa inoltre si deve concretamente impegnare nella gestione del gran numero di rifugiati, che sta drammaticamente aumentando nei Paesi confinanti con la Siria. In Turchia, Libano e Giordania sta crescendo il numero di siriani che sono fuggiti dalla guerra e che necessitano di assistenza. Nelle conclusioni della Conferenza interparlamentare di Vilnius della settimana scorsa, già citata, si è espressa esplicitamente la necessità e l'urgenza di un maggiore impegno europeo in questa crisi umanitaria. Rischia di essere comunque un vuoto appello, purtroppo; più efficace e concreto sarebbe un analogo impegno a livello intergovernativo degli Stati europei. L'Italia deve con forza richiedere a tutti gli Stati europei, non ai soli quattro

Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, i senatori del nostro Gruppo hanno molto apprezzato la chiarezza ed il coraggio con il quale oggi pomeriggio in quest'Aula il Presidente del Consiglio italiano ha definito, senza sfumature, odioso crimine contro l'umanità, che esige sanzioni durissime e immediate, il ricorso ad armi chimiche. Tanto più intelligente e coraggiosa questa definizione, in quanto accompagnata dalla precisazione, già definitasi - lo ricordava molto bene il collega Casini - nell'ultima settimana di agosto nelle Commissioni parlamentari, di un'Italia che continuava a dare speranza, credito e spazio alla legittimità delle Nazioni Unite senza partecipare a questa azione, al momento forse più di rappresaglia che di sanzione.

delle prospettive di non immediato ricorso alla sanzione o rappresaglia americana che sia. Questo però significa che smantellare l'arsenale siriano di armi chimiche farebbe diplomaticamente, politicamente e moralmente, sull'Assemblea delle Nazioni Unite responsabilità enormi. enormi. Ha ragione il presidente Letta quando definiva in qualche modo il dramma siriano quello di una «guerra per procura». Qui posso richiamare anche una considerazione del collega Casini: che cosa sono state le primavere arabe se non l'estrema dissoluzione di ogni sembianza di statualità di questi Paesi? Tra questi Paesi, la Siria, per usare il vecchio linguaggio reaganiano, era lo Stato canaglia per antonomasia, al quale abbiamo consentito che in questi anni si opponesse un'opposizione non meno canagliesca. non meno canagliesca. Già, ma se è così, se la contabilità delle vittime in questi due anni è quella che è e se c'è una contabilità di rifugiati impressionante (2 milioni di profughi che si accalcano ai confini di Libano, Giordania e Turchia), allora vuol dire che in questa guerra per procura l'obiettivo immediato può essere il già difficile smantellamento chimico della Siria. Ma, in prospettiva, non può non esserci lo smantellamento del nucleare iraniano. Perché un sistema per procura canagliesco, tra *Hetzbollah*, Siria e Iran, è vistoso ed evidente. speriamo che il segnale russo venga recepito (gli americani lo hanno già fatto) e - soprattutto - speriamo che sul territorio siriano le Nazioni Unite siano in grado di attivare i controlli, dobbiamo anche constatare come in questi anni abbiamo vissuto il fallimento istituzionale delle Nazioni Unite come istituzione di legittimità internazionale. Certo, siamo democratici europei che continuano a sperare, fin dai giorni dell'immediato dopoguerra, in questa grande idea delle Nazioni Unite, ma non possiamo tacere, proprio per le ragioni che affioravano nelle parole del collega Casini, a proposito di un Paese che è caro ad ogni europeo: Israele.

Cito il Capo dello Stato, senza intento di appropriarmene, ricordando che, con grande nobiltà, Giorgio Napolitano disse: «C'è un'odiosa forma di antisemitismo mimetizzato come antisionismo ed è quasi ovunque nel mondo targata Nazioni Unite». Ciò nonostante, non possiamo non guardare con interesse a quello che potrebbe dipanarsi sul filo della vicenda russa e americana e forse, senza nessun nazionalismo, che sarebbe provinciale, sulla base di qualche buona idea italiana, a San Pietroburgo. Infatti, il ruolo fallimentare dell'ONU sta anche nel problema che è già davanti a noi: i profughi. Se c'è un settore di fallimento è proprio l'assistenza ai profughi. In cinquant'anni la cultura, la burocrazia e la procedura delle Nazioni Uniti sono servite ad alimentare rancore nei profughi, ma mai ad assisterli nelle diverse realtà territoriali. Anche nella sua moderata quantità di risorse, il fatto che fra San Pietroburgo e Vilnius si siano trovate risorse importanti può essere un significato abbastanza incoraggiante per un ruolo europeo più incisivo. Tuttavia, non ci dimentichiamo - con questo concludo - che gli Stati Uniti d'America, non meno

La Costituzione, che lei sicuramente conosce, all'articolo 11 dice chiaramente che l'Italia è uno Stato che «ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». è andato al Vertice G20 portando la posizione dell'Italia, non ritenendo opportuno venire a discutere nelle Camere di questa eventuale partecipazione, ha voluto fare da solo: questo mi fa un po' paura. «Un odioso crimine contro l'umanità»: così è stato definito l'utilizzo delle armi chimiche

Queste armi convenzionali, signor presidente Letta, da chi sono fornite? Quali Nazioni forniscono e hanno fornito in questi anni armi alla Siria?

che ci fosse anche il Vaticano dietro a una delle aziende più grosse di armi nazionali. Non vorrei, signor Presidente del Consiglio, che la persona con cui ha parlato - ovvero Obama, premio Nobel per la pace

La guerra di Libia! Si ricordi dei danni che avete fatto in Sicilia, per i miei e per i suoi figli, signor presidente Letta. No alla guerra!

mi associo volentieri a chi l'ha ringraziata per aver scelto anche il Senato, oltre alla Camera dei deputati, per riferire sugli esiti del Vertice G20 di San Pietroburgo. Sono le cose non scontate, che in questo caso segnalano la centralità del Parlamento italiano, come previsto dalla nostra Costituzione, e che danno un segno decisamente positivo all'aver scelto questa strada.

è la ragione per la quale ogni iniziativa che va nella direzione di provocare minacce per la stabilità del Governo e per la governabilità, che lei rappresenta, va messa nella condizione di non provocare nessuna forzatura rispetto alle ragioni che hanno ispirato il suo programma di Governo. Infatti, un programma di Governo è fatto di tre fattori. Vi sono naturalmente i contenuti programmatici, ma vi sono anche due contenuti che stanno ai margini del programma, che sono però decisamente superiori: essi sono dati dalla credibilità interna e internazionale

Lo faccio perché condivido la posizione non scontata che l'Italia ha tenuto nel Vertice di San Pietroburgo e perché pare prevalga la via della ragione. Vi sono però tre questioni che l'Assemblea (e questa è una delle prime occasioni) deve affrontare, perché sono tre questioni nuove che io immagino, purtroppo, durevoli, che emergeranno ogni qual volta discuteremo di vicende e di relazioni internazionali. La prima riguarda la tenuta, la credibilità e l'efficacia degli organismi internazionali. Noi ci appelliamo spesso (e lo ha fatto anche lei) alle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite nascono alla fine della Seconda guerra mondiale in un quadro completamente diverso, naturalmente, rispetto a quello attuale e nascono per regolamentare i conflitti tra gli Stati: nascono per regolamentare i conflitti tra gli Stati: solo per questo scopo. Nascono infatti in un tempo che aveva visto la fine di due conflitti mondiali, a distanza di due decenni l'uno dall'altro. La domanda che le rivolgo e che rivolgo a me stesso è se un organismo di questa natura sia nella condizione, ancora oggi, di regolamentare conflitti che rarissimamente sono di uno Stato contro un altro Stato e che sempre più spesso prendono invece la dimensione di guerre civili: guerre civili in Paesi asiatici, in Paesi mediorientali, in Paesi africani e due guerre

conflitti non siano validi per regolamentare le guerre civili. Non ho obiezioni da sollevare circa il digiuno a cui ci ha invitato Papa Francesco,

gli Stati e le politiche hanno il dovere di agire, di prendere posizione, di intervenire non solo perché c'è una minaccia delle armi chimiche. Quando si ammazzano i civili nelle guerre civili, non c'è differenza tra l'uso di armi chimiche

Addirittura la Chiesa tenne, nel XII secolo, un Concilio per bandire l'uso della balestra, che era considerata un'arma poco onorevole, perché consentiva di uccidere a distanza, senza vedere il nemico in faccia. Anche l'arma chimica rientra in questa teoria, ma se le guerre da guerre fra Stati diventano guerre civili, noi abbiamo il dovere di dare una rappresentazione etica, istituzionale e politica a questa dimensione, creando gli strumenti perché gli Stati intervengano, soprattutto con la diplomazia. Quando si ammazzano i bambini, non c'è differenza fra un'arma chimica ed un kalashnikov: si ammazzano popolazioni civili e basta. La seconda questione, infine, riguarda l'Europa. L'Europa non ha ruolo e nell'assenza dell'Europa (e io la ringrazio per questo) ha trovato un ruolo ed una funzione l'Italia. Nell'Europa assente avrà un ruolo sempre maggiore la Russia imperiale ed avrà ai nostri confini, in Africa e Medio Oriente, un ruolo completamente nuovo la Cina. Tolto il Sud Africa e tolto il Medio Oriente (i Paesi rivieraschi e mediterranei), ormai ovunque i grandi investimenti appartengono a portafogli cinesi pubblici e privati. Senza Europa - vale quanto affermò di un grande giornalista, Montanelli, che disse che l'Europa era finita nel momento in cui i mercanti scelsero di comprarsi un blasone e diventare latifondisti e diventare latifondisti - sempre di più singoli Stati e, tra i singoli Stati, quelli che hanno più forza militare ed economica si sostituiranno agli organismi internazionali condivisi, come l'Unione europea. L'ultima questione riguarda la politica estera italiana. Ripeto: condivido e al suo posto avrei sottoscritto lo stesso documento che lei ha condiviso, ma abbiamo il dovere di valutare come maturano e come cambiano le cose. Nel Mediterraneo non è più centrale la questione israelo-palestinese; lo è stata per quarant'anni, ma non è lo è più. Il Mediterraneo è ormai il mare dei migranti, delle primavere arabe che sono tornate ad essere troppo rapidamente inverni, dei fondamentalismi religiosi e delle dittature laiche e teocratiche. Questo è il Mediterraneo. Noi abbiamo un doppio dovere. Lei sostiene giustamente Ginevra 2; io mi permetto di aggiungere, in conclusione, due altri elementi. apra il Governo una partita vera verso la Turchia. La Turchia è Mediterraneo ed è Europa, e non possiamo consegnarla a nessuna forma di estremismo. elemento questione è un'Italia che si faccia protagonista e chieda una Conferenza euromediterranea: non ricordo più da quanti anni manchi da un'agenda. già un luogo: potrebbe essere Erice, in Sicilia, per la sua tradizione contemporanea ed antica. Ma soprattutto c'è un'iniziativa che l'Italia deve assumere, perché senza Mediterraneo non esistono partite

- strumenti e operazioni, soprattutto per quanto riguarda le scelte sullo sviluppo, che sono di ben altra portata rispetto a quelle che abbiamo visto

Non vediamo scelte che indichino la possibilità di una ripresa forte dell'occupazione e, quindi, un sostegno forte alla domanda. Vediamo con preoccupazione continuare a crescere le disuguaglianze e la povertà nel nostro Paese.

un esempio di come non si facciano scelte sagge e, anzi, addirittura di come si vada a tagliare nei settori che potrebbero rappresentare una possibilità di sviluppo nel nostro Paese. Arriviamo ai temi che ci stanno e sono stati particolarmente a cuore nel dibattito che fino ad ora i miei colleghi hanno svolto. Mi riferisco alla situazione drammatica della Siria. Noi in queste ore siamo incoraggiati ‑ non è soltanto una speranza, perché le speranze bisogna poi coltivarle con le azioni concrete

chimici devono farci sperare con forza nella riapertura di uno spiraglio per evitare un'*escalation* militare. Noi abbiamo molto apprezzato

in maniera netta e inequivocabile contro un'eventuale azione militare, essendo ben cosciente - come ha ricordato il presidente Casini, di cui condivido in pieno l'intervento - dei pericoli - dei pericoli di un'azione militare all'interno della Siria. È evidente a tutti ormai, Presidente, lo sappiamo, che non si può certamente rappresentare la tragedia siriana come

sui ribelli. Mentre vediamo e abbiamo visto in questi mesi e anni crescere sempre più la forza e la prevalenza egemonica di tutte le formazioni jihadiste nel movimento dei ribelli, sappiamo che esistono associazioni movimenti che hanno un altro profilo, che sono di natura certamente molto più democratica e laica e che sono oggi completamente strette nello scontro tra Assad e i ribelli, che

Torno a ripetere: così come abbiamo apprezzato la posizione della ministro Bonino, riteniamo che il Governo italiano debba

una posizione che è stata condivisa da tutte le forze politiche e che deve essere lo strumento che l'Italia deve adoperare, in Europa e a livello internazionale, per

ed essere in modo chiaro, inequivocabile e senza ripensamenti contro una azione militare. Siamo stati molto aiutati, anche negli spiragli che si intravedono in queste ore, dall'azione (perché io così la definisco) del Papa, che non si è limitato semplicemente a convocare di preghiera collettiva sabato scorso, ma ha agito. Non solo egli ha saputo interpretare le coscienze, il volere e la sensibilità delle opinioni pubbliche internazionali (che stanno, per fortuna, pesando molto), ma il

Nessuno ha potuto farlo, perché si è tramutata in un'azione forte che ha richiamato le coscienze. Dobbiamo salutare anche il risveglio dei Parlamenti. Mi riferisco a quanto è accaduto in Gran

che intravede nello strumento negoziale l'unico strumento possibile in quell'area del Mediterraneo. *(Applausi Signor Presidente, colleghi senatori, onorevole Presidente del Consiglio, le comunicazioni dedicate ai risultati dell'atteso Vertice G20, svoltosi la scorsa settimana, giungono in un momento assai importante e delicato nel quale alle aspettative di una rapida uscita dalla recessione abbattutasi sull'economia internazionale si sono sommate le speranze di una soluzione al grave conflitto in Siria. L'ordine del giorno dei lavori, come è noto e come risulta dalle dichiarazioni rese a caldo proprio a San Pietroburgo dai Capi di Stato e di Governo partecipanti al Vertice,

ha dato certamente dei frutti sotto il profilo economico, ma questi sono assai circoscritti sul piano politico. Il G20 non è riuscito a trovare alcuna via d'uscita alla crisi determinata dall'uso delle armi chimiche lo scorso 21 agosto alla periferia orientale di Damasco. Come Gruppo Lega Nord, ci limiteremo oggi ad esprimere alcune semplici osservazioni. La prima è inesorabilmente una riflessione sul ruolo di questo nuovo *Forum* multilaterale, il cui peso nella *governance* mondiale è cresciuto parallelamente allo sviluppo delle economie emergenti, anche se con esiti finora piuttosto deludenti. Vogliamo dirlo chiaramente: il G20 non ci entusiasma. Infatti, mentre il vecchio G7 funzionava egregiamente nel coordinare le politiche economiche delle maggiori potenze occidentali, stabilendo di volta in volta su chi incombesse il compito di trainare l'economia internazionale, nel G20 le cose paiono andare molto diversamente. Lo si è attivato per provare a superare la crisi abbattutasi sulle maggiori economie occidentali coinvolgendo i Paesi emergenti. Non si è però riusciti nell'intento, anche perché i BRICS hanno cercato di sfruttare il momento per migliorare la propria posizione nel sistema internazionale. Lo schema pare ripetersi anche sul terreno politico-strategico, nel quale la sensazione è che le cose stiano andando persino peggio, in ragione della minore omogeneità geopolitica del raggruppamento. Riconosciamo che a San Pietroburgo sono uscite fuori cose interessanti, specialmente sotto il profilo delle misure da adottare per cercare di favorire una ripresa che sia accompagnata dalla creazione di posti di lavoro. È stato trattato il problema della gestione dell'indebitamento accumulato dagli Stati in questi anni difficili di rallentamento dell'economia e di crescita della disoccupazione, ma accordi veri sono stati raggiunti soltanto su aspetti del tutto secondari della vicenda economica contemporanea, quelli sui quali è più facile aggregare il consenso, come la lotta allo *shadow banking* (di cui ha parlato anche lei), alla finanza alternativa, ai fondi speculativi e ai titoli tossici. Non a caso, vi è chi, con riguardo al G20, parla ormai di un minilateralismo. Si è cercato in un certo senso, ancora una volta, di fare della manutenzione alla globalizzazione, enfatizzando, ad esempio, la necessità di continuare a garantire l'apertura dei mercati e il carattere unitario del mercato globale. Non si è però chiarito come questo obiettivo possa conciliarsi con l'evidente tendenza ad allestire raggruppamenti regionali più o meno allargati, dei quali l'Unione europea è l'esempio più evidente, ma non l'unico. soprattutto, sono rimaste fuori dalle discussioni - per quanto se ne sappia - sia il *tapering* (che è la riduzione graduale dell'immissione monetaria, all'orizzonte degli Stati Uniti) che gli ambiziosi progetti che concernono le aree transoceaniche di libero scambio (in futuro dell'area transatlantica dovremmo essere parte anche noi se andranno in porto i negoziati iniziati l'8 luglio). Il *tapering* è una novità importante perché, se verrà confermato, la Federal Reserve americana finirà presto (forse all'indomani delle imminenti elezioni tedesche) di iniettare i grandi quantitativi di dollari con cui ha alimentato l'avvio della ripresa negli Stati Uniti tenendo a galla tutto il sistema internazionale. Si tratta di ben 85 miliardi di dollari al mese che spariranno, alimentando verosimilmente una crescita dei tassi in America e forse un deflusso dei capitali dall'Europa. Paesi emergenti temono questo sviluppo, che avrà conseguenze anche da noi, nell'Unione europea ed ovviamente in Italia, sia che la Banca centrale europea (BCE) mantenga l'attuale indirizzo di politica economica monetaria, probabilmente svalutando l'euro, sia invece che decida di distaccarsene. Vedremo. Questo sarebbe stato il tema caldo: un tema che ci interessa notevolmente dal momento che, se si decidesse di alzare i tassi anche in Europa, per noi sarebbero grossi guai che dovremo cercare di affrontare. Sul piano politico-strategico, la corsa all'attacco in Siria, che fortunatamente adesso sembra rallentare, ha invece rivelato due spaccature profonde, sulle quali non è possibile tacere, dal momento che hanno influenzato anche la condotta del nostro Governo: è quella che ha condotto alla polarizzazione tra potenze del vecchio G7 e i BRICS, dei quali per una volta la Russia ha assunto la *leadership;* l'altra è quella che concerne l'Unione europea. Sotto il primo profilo dobbiamo rilevare, signor Presidente del Consiglio, una certa ambiguità di fondo, perché nel secondo giorno di lavori il nostro Governo è riuscito a figurare sia nell'elenco dei Paesi vicini alla Russia, nel respingere l'uso della forza contro la Siria, sia in quello degli Stati disposti a sostenere politicamente gli Stati Uniti nella loro azione punitiva anche in assenza di un mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. In questo caso apponendo una firma in calce a un testo scritto assai esplicito. Proprio questa scelta, che ci ha diviso dalla Germania, è valsa al suo Governo le critiche della cancelliera Merkel. E qui veniamo al secondo profilo che ho lamentato: la nuova frantumazione della solidarietà europea, solo in parte riuscita. In pratica, a San Pietroburgo il nostro Governo è riuscito a generare dubbi sulla nostra posizione (di fatto ambigua) di Paese che appoggia il ricorso alla forza, ma non vi si unisce, lanciando segnali incoerenti. La platea internazionale fatica a comprendere anche quando si fa riferimento a ostacoli costituzionali, che pure esistono, e che sono veramente e seriamente un margine invalicabile. Poco male, potremmo dire. In fondo non c'è nulla di nuovo, giacché in questa circostanza il Governo altro non ha fatto che muoversi nel solco di una consolidata tradizione del nostro Stato unitario, sempre pronto a pendolare da un lato all'altro dei maggiori schieramenti e debole nella difesa delle proprie visioni e degli interessi nazionali del Paese, anche le poche volte che è coerente Il fatto è però che di queste alchimie e indecisioni, trucchi e trucchetti escogitati per compiacere l'alleato americano, senza troppo urtare la Santa Sede, vi è chi può essere chiamato a pagare un prezzo elevato. E noi pensiamo oggi in particolare, signor Presidente, ai nostri soldati in Libano, che in caso di un conflitto con Damasco potrebbero rapidamente trovarsi ostaggio degli *hezbollah* proprio in ragione dell'appoggio politico a Washington. Per questo facciamo sommessamente notare come, prima di cambiare posizione in *dossier* tanto delicati, signor Presidente del Consiglio, sia opportuno cautelarsi adeguatamente riducendo rischi e vulnerabilità, evitando che debba provvedervi poi alla chetichella il suo Ministro della difesa che digiuna in piazza San Pietro, ma al tempo stesso manda il cacciatorpediniere Andrea Doria a proteggere, non si sa quanto efficacemente, i nostri caschi blu In conclusione, le chiediamo pertanto una minore approssimazione e una maggiore aderenza agli indirizzi annunciati appena lo scorso 27 agosto qui in Senato dal suo Ministro degli esteri. Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, parto dal documento che è stato firmato un documento che è stato pochissimo diffuso. Sono riuscito a trovarne soltanto una copia in inglese vorrei leggervene un piccolo passo da me tradotto: i firmatari hanno dato al Consiglio di sicurezza dell'ONU la responsabilità di condurre una risposta internazionale, ma concordano sul fatto che il Consiglio di sicurezza rimane paralizzato, com'è stato per due anni e mezzo. Il mondo non può attendere fallimentari processi che possono soltanto portare a incrementare la sofferenza in Siria e l'instabilità regionale. Beh, signor Presidente, questo non è affatto centralità dell'ONU: questa è una chiara delegittimazione dell'ONU! È un attacco alla paralisi del Consiglio di sicurezza che serve solo a giustificare Obama per una offensiva senza risoluzioni dell'ONU e per presentarsi al Congresso dicendo: guardate quante quante Nazioni sono con me favorevoli all'attacco. Questo documento firmato da 11 Nazioni, quattro delle quali europee, non è solo una condanna dell'uso delle armi chimiche, non è neanche solo un'attribuzione frettolosa della responsabilità dell'uso delle armi chimiche al Governo siriano: è una delegittimazione dell'ONU. Ciò è in contrasto assoluto con le dichiarazioni del ministro Bonino, peraltro reticenti, perché dice: no, si attacca solo con l'ONU, però non riferisce cosa l'Italia dice all'ONU di fare. fare. Rimane comunque il contrasto e addirittura rende ambigua persino la partecipazione del ministro Mauro a quella sincera iniziativa di Papa Francesco di una veglia per la pace. Non capisco cosa abbia pregato il ministro Mauro se il suo Presidente del Consiglio va a firmare un documento che dice chiaramente del Consiglio, penso che lei debba prendersi la responsabilità di dire cosa veramente vuole fare l'Italia e non parlare in maniera pacifista qui dentro e poi, di fatto, a livello internazionale avallare un attacco,

inoltre che noi abbiamo un contingente in Libano e, se ci fosse un attacco, sarebbe molto difficile che questo nostro contingente non venisse in alcun modo coinvolto nell'inevitabile allargamento allargamento del conflitto intorno alla Siria. Per questo motivo sono assolutamente in disaccordo con quello che ha dichiarato lei: non è vero che c'è un rapporto trasparente con il nostro Parlamento e non è vero che state perseguendo la centralità dell'ONU. Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il Presidente del Consiglio per averci relazionato su questo G20 complesso e articolato su due grandi emergenze: una largamente presente nel documento finale, l'altra invece prevalente nel dibattito. La prima, ovviamente, è la crescita economica e gli strumenti per garantire il superamento dell'attuale congiuntura economica mondiale, che è stato un tema prioritario fissato dalla presidenza russa. La seconda è la crisi siriana, sulla quale lei, Presidente, si è lungamente soffermato. Un importante approfondimento è rappresentato sicuramente 114 punti della dichiarazione finale e dai documenti allegati, in particolar modo il Piano d'azione di San Pietroburgo per la crescita e l'occupazione, che punta soprattutto agli investimenti. Temi su cui trovare una posizione condivisa: ritengo non sia stato facile per le grandi differenze fra i Paesi coinvolti in termini di struttura economico-produttiva, ma anche e soprattutto per i differenti livelli e gradi di ripresa della crisi. L'importanza di una convergenza su comuni posizioni risulta quindi ancora maggiore. Mi riferisco soprattutto all'impegno a definire una regolamentazione finanziaria per contrastare la frammentazione - lei l'ha citata nella relazione e il ritardo nella realizzazione di un'effettiva unione bancaria. La prospettiva G20 ha sicuramente riportato nuovamente la crisi dell'Italia nella più corretta dinamica internazionale. Questo non ci consente di nasconderci dai problemi specifici del nostro Paese e del nostro sistema economico e produttivo, ma ci permette di inquadrare i processi di causa ed effetto e di regolare, quindi, la nostra azione politica. Bene, dunque, gli impegni assunti dal nostro Paese sul taglio del cuneo fiscale, sulla riforma del mercato del lavoro, sul pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni alle imprese entro il 2014 e sulla semplificazione della giustizia amministrativa e civile. Mi soffermo adesso sulla questione che è stata poco presente nel documento finale del G20, anche per il mancato - mi sembra - raggiungimento di una posizione comune: la crisi siriana. Eschilo diceva: «In guerra la prima vittima è la verità». Quando non vi è un fronte e la guerra è così incivile da chiamarsi civile; quando gli scontri sono su base etnica e religiosa; quando non tutti combattono per la propria terra, è quasi impossibile discernere i buoni dai cattivi. La riflessione di Massimo Nava su «Il Corriere della Sera» di oggi porta ad una conseguenza: non si possono solo stilare delle graduatorie fra i buoni e i cattivi. È ciò che accade ormai da due anni in Siria. È ciò che accade in Medio Oriente da molto più tempo. L'Occidente, di fronte alla dicotomia, più esogena che endogena, fra sunniti e sciiti, si è schierato tendenzialmente dalla parte dei sunniti (con l'eccezione da tutti ricordata di Saddam Hussein), incorrendo - a mio avviso - nell'errore e nell'illusione che in certi conflitti sia ancora possibile scegliere. Se da un lato, infatti, gli sciiti uniscono al fondamentalismo, inaccettabile per Stati laici come i nostri, una certa stabilità e una certa omogeneità di posizioni, i sunniti ricoprono un amplissimo spettro di interpretazione dell'Islam, dal più laico al terrorista fanatico, rendendo anche la posizione occidentale difficile da sostenere. Oggi, Presidente, è l'11 settembre, come ha ricordato prima il presidente Letta, ed è impossibile non pensare a quanto è accaduto dodici anni fa. La forza e l'invasività dell'attacco alle Torri gemelle ha cambiato la nostra vita e tutt'oggi condiziona la nostra quotidianità. Ha portato allora e porta tutti noi ancora a dire «tolleranza zero». Ma la guerra in Iraq, i dieci anni di presenza in Afghanistan e le ultime primavere arabe ci mostrano che è difficile prendere anche solo posizione, se non comprendiamo appieno la complessità etnica e religiosa a cui ci troviamo di fronte. Le primavere arabe non hanno fatto che complicare questo già intricato quadro. La visione romantica a cui l'Occidente si è affezionato inizialmente si è trasformata in qualcosa di diverso, a seconda dei Paesi dove avveniva la rivoluzione. Nel riferire alle Commissioni esteri, il ministro Bonino ha fatto un passaggio fondamentale sulle diversificazioni interne al campo sunnita, diversificazioni che si stanno riflettendo anche sullo scenario siriano. Dobbiamo comprendere, quindi, che una fittizia dicotomia tra sunniti e sciiti non esaurisce l'analisi puntuale e rigorosa delle forze che si muovono sul campo,

La controversa attribuzione delle responsabilità dell'attacco con armi chimiche, le cui immagini hanno fatto il giro del mondo creando sgomento ed orrore, richiama quelle parole di Eschilo che ho cercato di riferire nella prima parte del mio ragionamento. Ma le immagini a cui siamo purtroppo abituati, di torture ed eccidi di massa da ambo le parti, non sono meno gravi fin dall'inizio di questa rivoluzione che ha tradito un po' tutti, parafrasando le parole pronunciate da Domenico Quirico all'atto della sua liberazione. In questi giorni, poi, due sono le notizie arrivate da quei luoghi: una buona e una pessima. La liberazione di Domenico Quirico è quella evidentemente buona. La caduta di Maaloula è quella sinceramente ed effettivamente molto cattiva. Se anche un laico come me può riconoscersi in alcuni luoghi indimenticabili della cultura cristiana, la caduta in mano a bande islamiste, qaediste e probabilmente criminali di Maaloula,

Una comunità che vive e ha vissuto in pace per duemila anni in quel villaggio viene spazzata via. Papa Francesco ha richiamato tutti - alla preghiera i religiosi, alla riflessione i laici - contro questa guerra. La posizione italiana, Presidente, è stata giustamente, fin dall'inizio, di condanna della violenza, come correttamente ha ribadito, ma di forte volontà di ricercare una soluzione diplomatica e politica. La richiesta di consegna delle armi chimiche da parte del regime di Assad, promossa dalla Russia, può andare in questo senso ed è giusto che sia discussa seriamente dalla comunità internazionale. Bene la proposta di Stati Uniti e Russia di una Ginevra 2, che è il luogo più adatto dove finalmente sia possibile avviare una riflessione autentica e condividere il concetto che oggi sia impossibile bombardare indiscriminatamente una delle due parti e lasciare campo libero a milizie alle volte islamiste, alle volte qaediste, alle volte criminali e che l'alternativa ad un regime assolutista, chiuso e dittatoriale come quello di Assad non possono essere califfati o regimi fondamentalisti. Troppi errori ha fatto, nel recente passato, l'Occidente nel Medio Oriente. Troppe volte, signor Presidente, abbiamo immaginato di esportare la democrazia e ci siamo trovati di fronte ai peggiori integralismi.

Concordiamo con le preoccupazioni, ma anche con le speranze che sono contenute nella sua relazione. Per quanto riguarda il suo intervento, vorrei sottolineare innanzitutto un aspetto interessante.

ma anche perché così si evidenzia meglio il nesso che esiste tra pace e sicurezza, da una parte, e sviluppo, dall'altra, tra diritti e legalità internazionale e possibilità della crescita, che è il nostro obiettivo. Quindi, ho apprezzato questo accostamento. Nel merito della prima parte del suo intervento voglio dire che noi consideriamo positivi i risultati ottenuti sui sette punti e sulle sette priorità avanzate dal nostro Paese, in particolare i risultati che abbiamo ottenuto sul terreno della crescita, del lavoro, della lealtà fiscale e della trasparenza. Mi sembra ne emerga una *road map* - per usare questo termine - una strada davanti a noi che è giusto portare avanti con determinazione. Sono anche dell'opinione che su tutta questa prima parte sarà utile ed opportuno tornare periodicamente in quest'Aula, tornare davanti al Parlamento, per misurare i passi avanti che otteniamo. Ne avremo occasioni negli in calendario sulla legge di stabilità e sui grandi provvedimenti; però penso che ogni tanto sia opportuno anche dare il giusto risalto a tutta la battaglia che stiamo facendo per la crescita, per il lavoro nonché per correggere l'impostazione europea di un'austerità a senso unico, che ha dato dei risultati, ma che bisogna anche temperare. Per quanto riguarda invece la questione siriana, sulla quale mi intrattengo un po' più a lungo, voglio dire che noi condividiamo le preoccupazioni e apprezziamo le scelte fatte fin qui dal Governo, e sottolineando quanto lei ha detto dal primo giorno, dal G20 di San Pietroburgo, fino ad adesso: è necessario avere ben chiara la comprensione della gravità e del rischio della situazione. Diciamo la verità: questa non è una crisi qualunque. Eppure non ci sono state e non ci sono ancora, anche nel sentimento comune dei nostri cittadini e della nostra popolazione, la giusta tensione e la giusta percezione della problematicità di questo passaggio. Ci sono tante cose dentro: dalla violazione dei diritti umani fino all'uso delle armi chimiche (ma giustamente anche quelle convenzionali vanno denunciate), senza dimenticare la drammatica situazione umanitaria che sta emergendo. del Consiglio, e io voglio semplicemente ribadirlo - l'esigenza di un forte impegno umanitario a favore dei profughi, soprattutto donne e bambini, che a centinaia di migliaia si vanno spostando e stanno aprendo un nuovo capitolo del dramma del Medio Oriente. Segnalo soltanto - perché è stato un tema di cui abbiamo parlato anche fra di noi - la drammatica situazione in cui si trova oggi il Kurdistan, che praticamente vede premere dalla Siria un esercito di persone, un fiume di persone che sta cercando riparo dalla guerra e dalle persecuzioni. C'è un'acutizzazione di tensioni e c'è anche una ricaduta negativa sull'economia che può avvenire: ecco qui, di nuovo, la connessione tra economia e sicurezza internazionale. Il tema è dunque molto serio,

tutti gli spazi a disposizione per la trattativa, per il negoziato, per una soluzione politica e per recuperare il giusto ruolo dell'ONU. C'è una proposta in campo, che è quella di mettere l'arsenale siriano sotto il controllo internazionale. Come è stato detto, organizzare una Ginevra 2 che rimetta in campo tutte le questioni del diritto internazionale. Facciamo tutti gli sforzi, anche nostri, per allargare questo spiraglio e ottenere i risultati sperati. Evitare i massacri, smantellare gli arsenali, ma anche isolare e sconfiggere le dittature e tutti i terrorismi che in questo momento si vanno presentando: questa è stata, sin dall'inizio, la posizione del suo Governo, Presidente del Consiglio, e noi l'abbiamo condivisa e sostenuta. La via maestra è quella dell'iniziativa politico-diplomatica. Non c'è spazio per un intervento militare senza l'avallo dell'ONU e senza un interlocutore chiaro ed affidabile, anche dopo l'esperienza drammatica dell'Iraq e le difficoltà che abbiamo vissuto nel caso libico. Quindi, la via politica è aperta, grazie anche all'iniziativa italiana. Questo dobbiamo dirlo: dobbiamo dare atto al Governo anche di un ruolo nuovo, più riconoscibile e più autonomo, senza con questo indebolire il rapporto con gli Stati Uniti e gli altri alleati. C'è stata una distinzione di posizioni sugli strumenti e non sugli obiettivi, non sugli ideali e sui valori di fondo da difendere. Comprendiamo anche le esigenze del presidente Obama quando parla di ideale di sicurezza e la sua denuncia degli orrori, che è anche la nostra. Presidente Letta, lei oggi ha detto che nei confronti del regime occorrono una condanna senza equivoci, una risposta e una pressione forte, continua ed adeguata. Su questo noi continueremo a sostenerla, perché condividiamo questa linea e questi sforzi. Mi avvio a concludere dicendo che, a nostro avviso, questo è il primo passo, quello che va fatto in questa fase per usare lo spazio negoziale che si è aperto, bloccare la guerra, salvare le vite e difendere gli spazi democratici. anche già guardare più avanti (lei, in qualche modo, lo ha detto). Questa vicenda siriana è destinata a rimescolare le cose, molti degli equilibri del Medio Oriente e del Mediterraneo e anche molte delle relazioni internazionali: dentro il mondo islamico, fra le grandi potenze e anche nella gerarchia delle diverse questioni presenti in quella zona e in quel territorio. Questo richiede di aver presente due nodi cruciali, su cui concludo. Il primo, aggirabile, è il tema del ruolo dell'Europa: se crediamo al multilateralismo, allora l'Europa deve esserci, compatta, attiva ed influente. Abbiamo preso atto con soddisfazione della segnalazione e dei passi avanti che sono stati compiuti anche a San Pietroburgo e dopo, però crediamo di poter dire che ancora non è sufficiente. Occorre un'iniziativa, una capacità unitaria dell'Europa che vincano anche le tattiche specifiche dei singoli Paesi. Questo è un grande problema, e credo che l'Italia possa svolgere un ruolo significativo. Infine, c'è il tema dell'importanza generale dell'area Medio Oriente-Mediterraneo negli equilibri generali, su cui esercitare un di più di capacità politica e diplomatica. Noi pensiamo che l'area del Medio Oriente e del Mediterraneo debba tornare ad essere il baricentro vero della politica europea, nel senso più lato. Specialmente nel momento in cui continuano ad andare avanti le tappe dell'allargamento, soprattutto a Nord e a Est, non dobbiamo dimenticare il valore fondante che ha per noi la frontiera del Medio Oriente, la frontiera del Mediterraneo, quella sulla quale l'Italia è maggiormente esposta. Per queste ragioni confidiamo che il lavoro del suo Governo su questi temi possa andare avanti fruttuosamente, non faremo mancare il nostro sostegno e crediamo che questi siano davvero gli elementi fondanti di una stagione politica che deve continuare a lavorare per dare tutti i suoi frutti.

ovviamente riteniamo che siano innanzitutto necessari una discussione e un approfondimento sul tema.

che è stato approvato in sede deliberante alla fine della scorsa legislatura, ma che consentisse una riflessione sul valore del sistema delle aree naturali protette, terrestri e marine.

di qualità per i nostri territori. Quindi, dopo vent'anni di applicazione della legge non possiamo che dire che il bilancio è stato assolutamente positivo. Vorrei ricordare in questa sede che nel nostro Paese si contano 23 parchi nazionali, 27 aree marine protette, 147 riserve naturali statali, circa 670 tra parchi e riserve naturali regionali, un totale di superficie terrestre protetta che supera i 3 milioni di ettari, per raggiungere i 6 milioni di ettari con le aree marine. Il sistema dei parchi ha fornito un contributo decisivo proprio sul fronte dello sviluppo qualitativo del nostro Paese: l'impulso al turismo naturalistico, a riscoprire i valori del territorio, le identità, il connubio che si è venuto sempre più a creare, per fortuna, con le produzioni agricole e agroalimentari di questi territori.

che hanno l'interesse prioritario nel conservare, nel mantenere e far fare un ulteriore salto di qualità a questo sistema, quindi nel senso migliore del termine. del termine.

del nostro disegno di legge - noi abbiamo cercato di evitare riportando tutti quanti a un tavolo, su una posizione comune, perché dobbiamo rimettere insieme le migliori energie per migliorare per migliorare l'assetto nonché il quadro legislativo e normativo. Quindi, il nostro sforzo è quello di trovare un punto di mediazione in senso alto per far sì che si possa effettivamente svolgere un lavoro proficuo. Le perplessità di alcune associazioni che sono state oggi nuovamente manifestate, per certi versi anche a ragione, sono relative

so che sono stati presentati altri disegni di legge di altri Gruppi parlamentari, quindi credo che noi dobbiamo fare di nuovo un lavoro che non dia

il fine delle aree protette. Le aree protette nascono per la conservazione degli ecosistemi, quindi non bisogna Non sto certamente parlando degli agricoltori, che anzi sono importanti e sono legati proprio alla finalità primaria della conservazione e della valorizzazione in senso buono.

e di valorizzazione di tutte le energie migliori che in questi anni hanno lavorato per il sistema delle aree protette del nostro Paese.

Federparchi, come ha già esplicitato anche in alcuni comunicati di questi giorni, ha assolutamente condiviso quel testo e ci sollecita ad intraprendere questo lavoro di

cattiva gestione di alcune specie invasive del territorio estremamente dannose per l'agricoltura. D'altronde, non ci troviamo qui oggi per discutere il merito

preferenziale al testo proposto. Mi meraviglia che chi dentro e fuori quest'Aula continua a tacciare il Parlamento di improduttività si opponga a procedure che invece consentono una discussione rapida e sicura del provvedimento. Il testo base, infatti, è assolutamente emendabile. Se qualcuno ha dalle proposte emendative, anche di larga parte del testo, le avanzi; ne discuteremo tranquillamente in questa sede, ma almeno arriveremo a un risultato, piuttosto che impantanarci in quello che è - questo che è - questo sì - un *iter* estremamente farraginoso che vede sempre protagonisti i disegni di legge di iniziativa parlamentare. vuol dare un segno di presenza e di attivismo per i suoi disegni di legge, oltre che essere sempre Camera di esame e ratifica dei decreti‑legge governativi, si utilizzino gli strumenti che il Regolamento mette disposizione: la procedura d'urgenza su un testo approvato nella precedente legislatura da uno dei due rami del Parlamento e solamente per poche settimane non trasformato in legge definitiva, perché già il testo aveva fatto un suo passaggio

un'espressione di giudizio positivo sull'intero testo, ma consente a quest'Aula di avere un testo base sul quale eventualmente apportare le modifiche che si riterranno necessarie.

Devo dare atto che nella passata legislatura è stato fatto un lavoro importante con una deliberazione unanime

ed è stata un buon provvedimento, come ricordava bene la senatrice De Petris. Sono nati i parchi, le aree protette marine

per il nostro Paese: luoghi dove si tutela la biodiversità e dove si sperimentano con successo nuovi modelli di sviluppo. Ricordo le lotte, per averle vissute personalmente, e lo scetticismo della politica e delle istituzioni. C'era un movimento culturale molto isolato nel 1991, ma alla fine è venuta fuori una buona legge. C'era scetticismo perché i parchi erano percepiti come enti inutili che ingessavano il territorio. Per anni c'è stata una battaglia, soprattutto culturale: una bottiglia che è stata vinta con i fatti, mettendo in cascina buon fieno. Adesso succede il contrario, colleghi senatori. Ho la percezione, anzi la convinzione che è mutata la condizione e la fase di osservazione che hanno avuto i parchi nel tempo. Ci sono benevole accettazioni da parte delle associazioni degli agricoltori; addirittura quelle venatorie comprendono l'utilità di avere aree protette. A tal proposito, è singolare l'azione di sostegno dei Comuni. Nella mia Regione c'è stato il tentativo di accorpare le aree protette e i parchi in un unico ente qualche anno prima avevano dimostrato ostracismo nei confronti delle aree parco, sono stati i primi a sostenerli e a difenderli. Credo che questa sia un'inversione dal punto di vista politico e culturale molto importante. Tutto questo è avvenuto grazie all'azione costante della Federparchi, che è un po' l'ANCI dei parchi, che ha saputo coinvolgere in uno spirito di leale collaborazione tutti gli enti e le istituzioni che hanno a che fare con le aree protette. Ha vinto, dunque, un modello di sviluppo che ha ancora margini di crescita. È per questo che alcuni accorgimenti normativi potranno facilitare ancora una maggiore espansione delle aree protette, una rottura dei propri confini, una contaminazione dei territori, esportando la qualità ambientale, paesaggistica e culturale, affinché questo patrimonio di tutti costituisca supporto a un nuovo modello di sviluppo. Questa è la sfida dei parchi per il futuro nostro e del nostro Paese: costruire alleanze con comunità locali, partecipando e guidando progetti di sviluppo locale sostenibile che abbiano al centro la natura, il paesaggio e la biodiversità. Il disegno di legge deliberato nella precedente legislatura dalla Commissione ambiente - sottolineo all'unanimità - unitamente agli altri disegni di legge di legge presentati da vari Gruppi devono essere la traccia per individuare un percorso comune e una soluzione unitaria che possa essere di aiuto al sistema. Quindi, senza contrapposizioni si dovrà trovare il modo di lavorare assieme sui testi che sono stati presentati e elaborarne uno condiviso uno condiviso che miri ad agevolare gli obiettivi sopra citati, ovvero continuare con la tutela ma anche agevolare forme di valorizzazione economica e sociale e semplificare le procedure.

Cominciamo a riportare i fari e la luce su un progetto importante, quello della valorizzazione del nostro patrimonio ambientale,

secondo luogo, noi vorremo aprire ‑ lo dirò in Commissione ambiente ‑ una fase d'ascolto e d'interlocuzione con tutti i portatori di interessi, partendo da chi ha avuto un ruolo fondamentale e straordinario, come le associazioni ambientaliste. essere nessuna preoccupazione quindi, perché credo si metterà in campo una strategia di ascolto e d'interlocuzione che ha dato risultati importanti. Infine, credo che non bisogna avere paura dell'innovazione; l'ho detto la settimana scorsa quando è stato approvato questo straordinario, secondo me, ordine del giorno sulla tutela e sulla difesa del territorio dal dissesto idrogeologico. Ho detto che la capacità riformatrice di un Paese si misura dal grado di attenzione che mette sulle questioni ambientali. alla stregua del lavoro che è stato svolto la settimana scorsa, ma anche qualche mese fa, su questioni importanti come l'Ilva, il Senato sarà ascoltare, saprà riflettere e decidere per il bene del nostro Paese. Con queste motivazioni, il Gruppo del Partito Democratico sostiene la procedura di urgenza per questo disegno di legge.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, ci troviamo a votare su questa dichiarazione di urgenza che viene dal passato: infatti, già nella scorsa legislatura si è arrivati

nell'estensione delle banchine portuali e dei retroporti. Una seconda causa è l'eccessivo costo del lavoro e dei servizi, che ha gravissime ripercussioni, soprattutto per i possibili investimenti stranieri. La terza causa è la lungaggine dei tempi per i controlli doganali, che porta il traffico marittimo, che passa

le pratiche in arrivo in modo più veloce. La nostra burocrazia, i nostri sistemi di controlli e di sdoganamento

con ricadute positive simili a quelle ottenute con la legge n. 84 del 1994, in grado di portare la nostra portualità a fare finalmente un salto decisivo e in positivo.

I rappresentanti del comparto hanno infatti chiesto audizioni in Commissione ed esprimono la necessità di una riflessione più approfondita sul testo, aprendo un confronto sul ruolo dei porti. Ovviamente la priorità è quella di scrivere una buona legge. Vanno bene dei tempi e l'urgenza, ma bisogna scrivere una buona legge, in grado di risolvere il più possibile le problematiche del settore e rilanciare le grandi potenzialità del nostro sistema marittimo, con indubbi vantaggi dal punto di vista economico ed ambientale. Condividiamo pertanto l'urgenza di una riforma portuale, a condizione però che in Commissione ci sia lo spazio per un ampio dibattito e per apportare le necessarie ed imprescindibili modifiche. scorsa legislatura il nostro Gruppo ha proposto degli emendamenti al testo, alcuni dei quali sono stati recepiti, ma altre e sostanziali modifiche sono rimaste inascoltate in questa sede sarebbe il caso di rifletterci e di riprenderle con più attenzione. Mi riferisco principalmente alla possibilità di assicurare una maggiore autonomia finanziaria ai porti e una maggiore liberalizzazione del lavoro nell'ambito degli stessi. Inoltre c'è il problema del congelamento delle concessioni, che potrebbe rappresentare un grave pericolo, perché le concessioni così lunghe - per noi eccessivamente lunghe - rischiano di ingessare una situazione che invece necessiterebbe di dinamismo, di dinamismo, di vivacità commerciale e imprenditoriale. Concludendo, riteniamo condivisibile la scelta di discutere al più presto questo provvedimento in Commissione, con un occhio però rivolto al regolamento europeo che fisserà le norme in tema di aiuti di Stato ai porti, trasparenza finanziaria e, più in generale, alle liberalizzazioni, e con un occhio rivolto alle esigenze del mondo portuale per aprire un dibattito serio e attento sul tema, che dia spazio a proposte di modifica tese ad attuare una vera e, finalmente, più efficace riforma del nostro sistema portuale. *(Applausi

Purtroppo non sempre ciò viene percepito dall'opinione pubblica e dalla maggior parte dei soggetti politici. Proprio il Governo Monti ha per la prima volta inserito l'autonomia finanziaria, anche se solo dell'1 è stato però un forte segnale al settore di attenzione e cambiamento. Bisogna rendersi conto che i porti generano un gettito fiscale molto importante per il Paese nel corso del 2011, i porti italiani hanno generato un gettito fiscale di 13 miliardi di euro) e che se non destiniamo una parte di questo gettito fiscale a opere che consentano al sistema portuale di adeguarsi agli standard mondiali, questo gettito diminuirà fortemente nei prossimi anni, ben al di là di quello che potrebbe essere l'aumento della percentuale dell'autonomia finanziaria. Si rischiano quindi di perdere, a vantaggio di altri Paesi europei: traffici, gettito fiscale e occupazione diretta e indiretta che ruota intorno al nostro sistema portuale. È molto importante quanto sta portando avanti il ministro dei trasporti Lupi, che dimostra una forte attenzione agli investimenti per migliorare e completare i corridoi di collegamento tra l'Italia e il Nord-Europa. Se però i Corridoi arriveranno in porti vecchi e inadeguati a ricevere le nuove navi, di dimensioni tali che non si potevano assolutamente immaginare sino a qualche anno fa e per le quali oggi non siamo assolutamente preparati, anche questi investimenti diventeranno totalmente inutili nei Corridoi. Noi abbiamo la necessità di spostare le dighe e di fare una serie di interventi. Ma che cosa chiede il sistema portuale italiano?

Credo sia auspicabile - questo sì - farlo anche per decreto-legge, perché è urgente, non si può aspettare. Il risultato non sarà che il Paese conserverà il restante 2 per cento se non vogliamo aumentarlo, bensì crollerà il gettito fiscale derivante dai traffici, di cui l'Italia, di anno in anno sempre più significativa. Sarebbe davvero un atteggiamento miope e dannoso. A parte questo aspetto fondamentale, facendo parte della Commissione trasporti, dove abbiamo dibattuto sulla posizione da prendere sulla riforma della legge n. 84 del 1994, ho espresso più volte le mie perplessità sul disegno di legge, avendo ascoltato diverse posizioni dei primari operatori e associazioni nazionali. Sono lieto che ieri in Commissione sia passata la mia richiesta di concedere alcune audizioni ai primari interlocutori nazionali, anche nel caso in cui oggi il Senato voti a Non sappiamo certo quanto tempo avrà questo Governo per portare avanti questo disegno di legge, ma certamente se si pensasse di ripartire da zero - come dicono alcuni - non credo che ci sarebbe alcuna possibilità di far vedere la luce alla riforma della legislazione sui porti di cui stiamo parlando. Viene da pensare che chi si schiera contro, di fatto, vorrebbe solo che restasse tutto come è oggi, visto che su questo disegno di legge possiamo comunque fare delle modifiche in via emendativa anche significative. Qui si inserisce un fatto che ritengo grave di questi giorni e che mi ha convinto ancora di più ad esprimere parere favorevole alla richiesta di urgenza: il grave comportamento adottato da alcuni membri della Camera dei Deputati, che stanno di fatto minacciando l'indipendenza e l'obiettività dei membri del Senato, in particolare di coloro i quali come me sono anche membri dell'8a Commissione, chiamata a esaminare i disegni di legge. Questa intromissione si è verificata già dalla fine di luglio, anche in forma pubblica attraverso gli organi di stampa, che riportano dichiarazioni di onorevoli che ritengono di dover avvisare (o dovrei forse usare il termine minacciare) che se in quest'Aula voteremo a favore dell'urgenza del disegno di legge loro l'affosseranno non appena arriverà alla Camera. Ritengo questo un comportamento assolutamente irrituale e irrispettoso delle istituzioni, oltre a violare di fatto il sistema bicamerale che a oggi regola il funzionamento del nostro Parlamento. Penso anche che dobbiamo estremo rispetto al lavoro fatto dai senatori della scorsa legislatura, che aveva portato ad approvare questo testo, anche se - ribadisco - dovremmo prima audire pochi e primari attori del settore per valutare come proporre emendamenti migliorativi già al Senato, in Commissione e in Aula. In tempi brevi potremo inviare alla Camera il disegno di legge, che a quel punto mi auguro, senza preconcetti e difesa di interessi di chicchessia, apporterà le modifiche che riterrà opportuno e non affosserà il come dichiarato da alcuni soggetti, non privi di interesse diretti nel settore, per rimandarlo in Senato per la terza lettura e approvazione. Ringrazio i colleghi della Commissione 8a, con i quali abbiamo lavorato molto bene, per il chiaro e sereno dibattito costruttivo,

Ci tengo però a precisare che una riforma della legislazione portuale formulata in un testo unitario che raccolga tutta la legislazione in materia, oltre che auspicabile, è veramente necessaria. Pur comprendendo la volontà dei firmatari di utilizzare la dichiarazione di urgenza ai sensi dell'articolo 81 del nostro Regolamento, non la condividiamo. Il provvedimento è urgente, anzi, meglio, è prioritario, proprio perché tanto atteso, ma una legge di questa entità deve essere al passo con i tempi, deve raccogliere i suggerimenti della maggior parte delle associazioni di categoria e di tutti quegli operatori ed enti che giorno per giorno trattano, sul campo, la materia. La trattazione d'urgenza non permette la necessaria e attenta trattazione e ci espone al rischio concreto di approvare un testo già sorpassato. Non ci permette quegli approfondimenti atti a valutare le disposizioni di legge promulgate in materia portuale.

Dello stesso avviso appaiono le associazioni di categoria che di recente hanno rilasciato dichiarazioni alle agenzie di stampa che supportano queste riflessioni. Infine, mi permetto di richiamare la centralità del Parlamento, perfetta sede, almeno a Costituzione vigente, dove dal confronto con le realtà del nostro Paese e dal confronto fra noi possono uscire leggi approfondite e a misura d'uomo che soddisfino sia le necessità del legislatore, che quelle degli operatori del settore, apportando benefìci a tutti i cittadini. Diamo quindi priorità alla trattazione del provvedimento nell'8a Commissione e favoriamone,

quindi tutti i passaggi per una procedura ordinaria. Unica garanzia di un confronto costruttivo è proprio la trattazione normale. Per tutti questi motivi il Movimento 5 Stelle voterà contro la **richiesta di adozione della

Presidente, ribadisco gli stessi concetti che ho espresso nell'annunciare il voto favorevole del Popolo della Libertà per il precedente disegno di legge.

Commissioni e poi dall'Assemblea, trasmesso alla Camera e non approvato, per poche settimane di tempo, in via definitiva. È vero che il tempo certamente è passato dall'approvazione di questo testo in Senato) ma è anche vero che ne sono passati venti dalla prima formulazione della legge di regolazione delle autorità portuali del nostro Paese. Quindi, abbiamo il dovere di procedere con la massima urgenza, e naturalmente anche con la massima razionalità, esaminando tutte le possibili modifiche a quel testo: ciò è previsto assolutamente dal Regolamento. Ribadisco anche in questa dichiarazione di voto che qui si tratta di promuovere una procedura e non di accogliere un testo preconfezionato. quindi convinto che, ancora una volta, anche in quest'occasione il Parlamento potrà dare buona prova di sé approvando un disegno di legge di iniziativa parlamentare - anche quello della della precedente legislatura lo era - cercando di superare le abituali farraginosità del nostro Regolamento che, come è dimostrato da ciò che oggi proponiamo, spesso nell'arco di una legislatura non consente di concludere

orgoglio, se mi è consentito il termine, da parte del Parlamento, delle sue prerogative e della sua volontà di legiferare e non solamente di ratificare provvedimenti governativi.

di saper legiferare e di saperlo fare nei tempi necessari per seguire le esigenze del Paese; esigenze concrete e reali degli operatori. Noi che viviamo le città di mare sappiamo benissimo che molto spesso le esigenze degli operatori sono diverse da quelle dei gestori, che talvolta talvolta sono proprio i protagonisti della resistenza alle riforme. Il vero conservatorismo molto spesso è più negli apparati intermedi tra la politica e gli operatori che non nelle Aule parlamentari. Noi speriamo, portando in porto questo disegno di legge, di confermare la mia intuizione - se la possiamo chiamare in questo modo - che noi vogliamo fare le riforme ma spesso è il Paese che si prodiga a bloccarle.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito Democratico condivide pienamente la richiesta di applicazione dell'articolo 81 del Regolamento alla riforma dell'ordinamento portuale, per diverse buone ragioni che mi appresto sommariamente ad elencare. In primo luogo, il fattore relativo al tempo necessario per approvare una legge non costituisce mai un aspetto secondario, specie quando l'attesa di riforma per l'attuale ordinamento rappresenta un'esigenza avvertita da tempo. In questo senso, voglio solo ricordare all'Aula che ad una revisione della legge n. 84 del 1994 si lavora in questo ramo del Parlamento, con diversi propositi ed alterni successi, da più di dieci anni, senza però mai arrivare ad una sua definitiva approvazione. In questo lasso di tempo sono intervenuti fattori di cambiamento nel settore dello *shipping* internazionale davvero considerevoli: da un incremento dimensionale delle flotte, che non ha precedenti nella storia della navigazione, ad un'innovazione nell'organizzazione della logistica delle merci, che ci ha visto rincorrere di volta in volta drastici fenomeni di *dumping* sociale, ambientale ed economico‑finanziario. In sostanza, si tratta di mutamenti tali da far ritenere il periodo che stiamo vivendo una fase di cambiamento davvero epocale. Basti pensare che, nei vent'anni che ci stanno alle spalle, il nostro Paese ha beneficiato in termini di incremento dei traffici grazie essenzialmente al suo posizionamento geografico che lo vede come sappiamo - naturalmente collocato al centro di un Mediterraneo rivitalizzato prevalentemente dai traffici provenienti dal *Far East* lungo la rotta Suez-Gibilterra. Per i prossimi dieci anni, però, sono previsti cambiamenti significativi persino sulle rotte dello *shipping* internazionale, tali da far prevedere una perdita effettiva di quella centralità ritrovata del Mar Mediterraneo a favore delle rotte atlantiche Sud-Sud, di quelle pacifiche e persino come abbiamo visto recentemente - di quelle polari, inaugurate anche dalle enormi navi rompighiaccio di fabbricazione asiatica. In questi scenari di cambiamento così enorme il nostro Paese si dibatte con una legge ordinamentale approvata sul finire della prima Repubblica che, per quanto abbia costituito abbia costituito un fattore di svolta e di cambiamento fondamentale positivo, è comunque precedente alla riforma del Titolo V della Parte II dellanostra Carta costituzionale, la quale ha visto sostanziali modifiche nel riparto delle competenze in questo settore. Va subito detto per correttezza che il testo di legge per cui viene richiesto l'esame con procedura abbreviata è probabilmente insufficiente a cogliere in maniera esaustiva tutte le novità

nell'auspicio definitivamente, una fase con le necessarie modifiche ordinamentali rese nel tempo ancor più stringenti dalla situazione di crisi economica. Il nostro sistema portuale ha bisogno innanzitutto di riconoscersi compiutamente nelle sue diverse vocazioni e specializzazioni esistenti e potenziali, recuperando una missione complessiva nel suo inquadramento e nella sua collocazione internazionale, e cercando nella conferma della sua natura essenzialmente pubblica, dovuta all'insistenza delle strutture di demanio marittimo negli ambiti portuali, la possibilità di conoscere e frequentare una maggiore dinamicità imprenditoriale, fattore essenziale per l'incremento dei traffici esistenti e per quelli di nuova acquisizione. Oltre la revisione dell'attuale ordinamento ritengo ci sia anche richiesto di aprire una fase di confronto capace di traguardare l'attuale situazione ai processi di cambiamento in atto che ho richiamato. Non sarà questo un dibattito da improvvisare né un lavoro facile né breve, anche per i cambiamenti culturali che probabilmente si renderanno necessari. Per questo - ritengo - è senz'altro meglio condurlo in una condizione in cui la situazione ordinamentale attuale venga almeno sanata dalle difficoltà e dalle contraddizioni esistenti, la prima delle quali è costituita dal sistema delle risorse disponibili, ma anche dalle norme di pianificazione e dai poteri riconosciuti negli ambiti portuali. Si tratta di aspetti essenziali, per i quali il disegno di legge in questione nasce e si articola, a partire da un'effettiva autonomia finanziaria per gli scali portuali (richiamata anche negli altri interventi), essenzialmente finalizzata alla realizzazione delle infrastrutture necessarie al loro ammodernamento, ma anche dalla necessità di più congrue norme di pianificazione, che consentano una maggiore semplicità delle operazioni di dragaggio per l'approfondimento dei fondali portuali, oggi - anche questo aspetto è stato fattore indispensabile per i nostri porti, al fine di essere scalati da navi di sempre maggiore stazza e, conseguentemente, di sempre maggiore pescaggio. Sono infine necessarie norme di pianificazione che consentano l'approvazione di piani regolatori o di loro varianti anticipatrici non più in tempi biblici e indefiniti, ma in tempi certi e ragionevoli, grazie a procedure chiuse e rigorosamente definite nelle titolarità e nei tempi di approvazione, fattore quest'ultimo indispensabile per poter consentire ipotetici investimenti di capitali stranieri interessati ai nostri scali come ha recentemente auspicato lo stesso Governo - anche per altri contesti infrastrutturali. Tutti aspetti, questi, adeguatamente definiti nel disegno di legge in questione e al tempo ‑ come diceva appunto il senatore D'Alì ‑ ampiamente condivisi dall'intero *cluster* portuale. In ultimo, non voglio sottacere due questioni che possono pregiudicare il lavoro a cui, con rinnovata lena, intendiamo apprestarci. *In* *primis*, la durata di questa legislatura, la cui previsione al momento non consente facili ottimismi e su cui però non possiamo dare niente per scontato. Forse, proprio per questa paradossale situazione, occorre sfruttare ogni possibilità e ogni contesto, per non rendere vano neppure un giorno di un Parlamento legittimamente eletto e nel pieno delle sue funzioni e delle sue prerogative fino al giorno del suo scioglimento. Infine, c'è il ruolo che in questo percorso ‑ che noi, come Senato, ancora una volta avviamo ‑ vorranno giocare l'altro ramo del Parlamento e il Governo. Per quanto riguarda la Camera, essendo credo superfluo richiamare la sua autonomia e le sue prerogative, mi auguro soltanto che, con le modifiche che riterrà massimamente più opportune, riesca a completare i propri lavori in tempo utile per una definitiva approvazione. Per quanto riguarda il Governo, anche in questa sede mi sento di ripetere quanto più volte affermato nel corso di questi mesi: faccia della legge ciò che vuole. Non ci sono atteggiamenti, in questo senso, di sterile primogenitura da parte di nessuno. Per quanto ci riguarda, ci sono norme che possono da subito essere assunte e tradotte in prossimi decreti‑legge:

e mai formalmente disconosciuti da nessuno dei soggetti interessati. Norme che potrebbero vedere la loro agevole ratifica in brevissimo tempo. In conclusione, la procedura abbreviata che prevediamo per l'esame della riforma dell'ordinamento portuale a nostro modo di vedere non costituisce quindi soltanto una possibilità che il Regolamento parlamentare ci consente, ma vuole essere in sé anche un segnale forte e chiaro, un messaggio sia alla comunità portuale italiana, che attende da anni maggiore concretezza e realizzazione dei nostri lavori, sia ai soggetti istituzionali chiamati ad interagire con l'*iter* di approvazione delle norme in questione. Riponiamo la nostra fiduciosa speranza affinché, nel rispetto delle prerogative e dell'autonomia di ciascuno, non si renda il meglio, inteso come le modifiche che verranno ritenute necessarie da apportare al testo, anche in quest'Aula, nemico del bene, inteso come l'effettiva approvazione di norme da troppo tempo attese per dare maggiore slancio all'economia marittimo‑portuale, settore economico e imprenditoriale strategico e fondamentale per il nostro Paese. *(Applausi

per informare quest'Aula che alcune norme sono state già recuperate all'interno dei decreti-legge convertiti in legge recentemente. Inoltre, il Ministero sta predisponendo un testo

accolte in alcuni provvedimenti e, per quanto riguarda le altre, c'è già un provvedimento *in itinere* che, a questo punto, mi auguro possa essere emanato sotto forma di decreto-legge e, quindi, possa avere gli stessi caratteri di rapidità. le norme di semplificazione ambientale contenute nel disegno di legge sono molto attese da molti comparti economici e soprattutto da parte del settore agricolo e di alcune comunità, come quelle delle piccole isole e di altre comunità comunità che possono meglio gestire il loro cosiddetto verde pubblico. Sono quindi disponibile al ritiro della richiesta di procedura d'urgenza e mi faccio carico, in questa disponibilità, dell'assenso degli altri colleghi che hanno firmato con me la richiesta. Sono certo che anche le altre forze politiche convengono sul fatto che un esame di un decreto-legge governativo possa essere sostitutivo anche di questa procedura con gli stessi termini, forse anche con tempi ancora più veloci di definitiva approvazione. Infatti, il decreto-legge deve fare il suo passaggio tra Camera e Senato in 60 giorni, mentre la procedura d'urgenza prevede un'immediata discussione del disegno di legge nel ramo del Parlamento che l'approva, però poi è rimessa anche alle valutazioni regolamentari dell'altra Camera e, quindi, potrebbe avere un *iter* ancora più lungo. Grazie, Grazie, penso che le precedenti votazioni in materia di urgenza abbiano interpretato assolutamente la volontà della stragrande maggioranza del Parlamento, ma anche di coloro che hanno manifestato alcune perplessità, perché la trattazione dei disegni di legge che abbiamo proposto all'attenzione del Parlamento con la procedura d'urgenza è sempre stata assolutamente condivisa da tutte le forze politiche. Non mi sarei permesso Grazie,

il senatore D'Alì ha ritirato la richiesta di procedura abbreviata per tutti i disegni di legge in oggetto, e quindi anche per

Essa illustra l'impatto stimato delle misure incluse nel decreto-legge n. 102 in esame alla Camera dei deputati e fornisce una prima analisi della situazione economica in vista della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF 2013. Ricordo che le misure previste nel decreto riguardano un ulteriore pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione rispetto a quelli già disposti dal disegno di legge n. 35 del 2013, il rifinanziamento della cassa integrazione guadagni, un'ulteriore salvaguardia dei lavoratori dall'innalzamento dei requisiti d'accesso al pensionamento, misure a sostegno delle famiglie su mutui per la prima casa ed affitti, nonché il riordino della tassazione sugli immobili. Il complesso delle nuove misure lascerà inalterato l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche riferendosi unicamente al fabbisogno finanziario finanziario e al debito. In merito alla situazione economica, la Relazione riporta la stima preliminare del prodotto interno lordo riferita al secondo trimestre, diffusa dall'ISTAT il 10 agosto, che registra una contrazione di 0,2 punti percentuali, migliore delle aspettative dei principali previsori, mentre per il dettaglio delle componenti del PIL rimanda alla nota sui dati di contabilità trimestrale che è stata diffusa ieri dall'ISTAT. La cosiddetta crescita acquisita fino a tutto il secondo trimestre del 2013 è indicata come pari a -1,7 maggiore di quella prevista nel quadro economico del DEF, pari a -1,3 per cento per l'intero anno, prevalentemente a causa del risultato negativo del primo trimestre e di alcune revisioni statistiche al profilo del PIL del 2012. Tuttavia, le ultime informazioni disponibili sembrano confermare, secondo il Governo, l'ipotesi avanzata nel DEF di una ripresa dell'attività economica nella seconda parte dell'anno. Va rilevato però che i conti economici trimestrali dell'ISTAT, al secondo trimestre 2013, certificano che la variazione acquisita per il 2013 è pari a -1,8 La Relazione sottolinea alcuni segnali favorevoli provenienti dal livello della produzione industriale, che ha interrotto la tendenza alla caduta nel secondo trimestre dell'anno, dagli ordinativi, inclusi quelli provenienti dall'interno, e dagli indicatori di fiducia. Queste tendenze iniziano a rafforzarsi e a estendersi dall'industria ad altri settori dell'economia. Gli indicatori di fiducia delle famiglie e l'andamento delle vendite al dettaglio prefigurano un miglioramento nella domanda interna nel suo complesso nel corso dei prossimi mesi, con effetti favorevoli sul settore dei servizi. Sono confortanti anche gli ultimi dati sulle esportazioni. L'andamento del credito all'economia, invece, fornisce ancora segnali contrastanti: la mancanza di un'adeguata espansione potrebbe costituire un fattore di rischio per le prospettive di ripresa. La valutazione dell'impatto sull'economia dell'ammontare aggiuntivo di pagamenti dei debiti per 7,2 miliardi di euro nel 2013 rispetto alla legislazione vigente (decreto-legge n. 35 del 2013) assume che la maggiore iniezione di liquidità nel 2013, se attuata in tempi sufficientemente rapidi, darà alle imprese benefici in termini di maggiori investimenti, produzione e consumi. Rispetto alla legislazione vigente, i pagamenti aggiuntivi dei debiti pregressi della pubblica amministrazione producono, secondo le stime del Governo,

Il miglioramento della crescita è principalmente riconducibile alla maggiore crescita degli investimenti e, in misura minore, dei consumi. Gli ulteriori pagamenti di debiti pregressi della pubblica amministrazione pari a 7,2 miliardi di euro

Tale maggiore debito pubblico sarà considerato nella valutazione del rispetto della regola del debito prevista dal *fiscal compact* e applicata all'Italia nel 2015 sui dati dei tre esercizi precedenti, che quindi includono anche il 2013.

Esso è stato considerato un aumento del debito pubblico dovuto ad un aggiustamento *stock*-flusso e la sua valutazione da parte del Consiglio europeo ai fini dell'applicazione della regola sul debito è assimilata ai cosiddetti fattori rilevanti. che appuri, perché va appurato, se tale debito pubblico aggiuntivo sia compatibile con il profilo di riduzione previsto dalla predetta regola (quella del *fiscal compact*). Ricordo che ci sono 7,2 miliardi aggiuntivi nel 2013. Il 2013 fa parte del triennio di riferimento

questo debito pubblico aggiuntivo è compatibile con il profilo di riduzione previsto dal *fiscal compact*. La cancellazione del pagamento della prima rata dell'IMU sull'abitazione principale di proprietà a decorrere dal 2013 ha effetti positivi sul reddito disponibile delle famiglie, liberando risorse che dovrebbero, almeno in parte, essere destinate ai consumi già dal 2013. L'insieme delle misure per il settore immobiliare contenute nei provvedimenti introdotti di recente dal Governo (anche non facenti parte del decreto-legge n. 102 del 2013, ma che costituiscono un insieme unico di iniziative per il settore immobiliare) si tradurrebbe in un aumento del PIL pari a 0,1 punti percentuali a partire dal 2013 riconducibile quasi esclusivamente agli investimenti. Per avere un analogo effetto negli anni successivi le misure adottate nel 2013 dovrebbero esser rese strutturali. A questo proposito, un punto essenziale è appurare se tale valutazione dell'effetto delle misure di sostegno al settore immobiliare sull'economia sia considerata al netto del presumibile effetto contrario esercitato dalle norme di copertura previste dal decreto-legge n. 102. Le nuove stime di finanza pubblica per gli anni 2013-2017 elaborate sulla base delle nuove previsioni di crescita dell'economia e dell'impatto delle misure contenute nel decreto-legge n. 102 mostrano un peggioramento dei valori programmatici di indebitamento netto della pubblica relativamente al solo biennio 2014-2015, mentre restano, viceversa, confermati gli obiettivi indicati nel DEF 2013 per gli anni 2016-2017. Sia il fabbisogno del settore statale sia il livello del debito pubblico aumentano di circa 8 miliardi di euro per effetto della nuova iniezione di liquidità prevista dal provvedimento di urgenza in questione. Alla copertura finanziaria del provvedimento si fa fronte attraverso maggiori entrate IVA (925 milioni) connesse al pagamento dei debiti commerciali, la definizione per 600 milioni di contenziosi nel settore dei giochi, l'acquisizione al bilancio di una quota delle entrate relative alla tariffa elettrica (300 milioni) e il ricorso a tagli di spesa per circa un miliardo. In relazione alla copertura di parte degli oneri del provvedimento mediante maggiore gettito IVA per circa 925 milioni di euro, connesso all'incremento del pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione per 7,2 miliardi, andrebbe chiarito il motivo della diversa quantificazione rispetto a quanto analogamente previsto n. 35 del 2013, allorché il maggior gettito IVA era di circa 600 milioni a fronte di un pagamento di debiti pregressi pari a 20 miliardi di euro. Chiedo al Governo una particolare attenzione riguardo a tale quesito, perché è evidente che, a seconda della stima che il Governo ritiene più corretta, possono prodursi eventualmente nuove risorse IVA per il pagamento dei debiti commerciali. Però, prima di considerare una misura di questo tipo, è utile una riflessione del Governo, non soltanto in questa sede, ma eventualmente anche per il prosieguo e soprattutto per la sessione di bilancio, per una quantificazione più esatta delle risorse provenienti dall'IVA. Si tratta di risorse considerevoli che, in un momento di coperture diciamo così, forse potrebbero essere di ausilio o forse no. In termini di bilancio dello Stato, le misure suddette determinano la necessità di ridefinire prudenzialmente il saldo netto da finanziare del 2013 in aumento

Ricordo che i tempi del dibattito sono stati ripartiti tra i Gruppi secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo. Le proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione.

che sono sentiti in modo più consistente dai *media* e dall'opinione pubblica, oggi sarebbe piena. Siccome si deve parlare di economia, della condizione di disastro nella quale versa questo Paese, di come uscirne e dare una valutazione sugli strumenti che ha posto in essere il Governo, bisogna quindi parlare della vita delle persone, di come riusciamo a consentire loro di avere un lavoro e un reddito, di potersi costituire in nucleo familiare, di poter avere una prospettiva per il futuro, l'Assemblea non è interessata e la presenza è ridotta. Ciò, perché noi abbiamo una gerarchia di valori che ci porta a riflettere spesso se siamo nel giusto o se sbagliamo.

non voglio soffermarmi sulle tendenze dell'economia. Come abbiamo già visto, siamo in recessione: alcuni dicono che è una recessione attenuata, altri dicono che è una recessione prolungata, ma rimane il fatto che siamo in recessione. Allora voglio tentare di fare una simulazione, così come fa questa Relazione, perché viviamo di stime, di ipotesi che prendiamo per buone senza aver fatto le necessarie verifiche. Si stima la crescita del PIL in ragione, per esempio, del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione verso le imprese, però non sappiamo se le imprese stanno incassando. Sappiamo che la pubblica amministrazione centrale forse ha trasferito alle pubbliche amministrazioni locali una parte della dotazione finanziaria che è stata stanziata

al quale rinunciamo e avessimo investito questo miliardo e mezzo di fiscalità che rimane nelle tasche, distribuite, di italiani più o meno facoltosi,

di euro in un grande piano di rilancio dell'edilizia, non avremmo avuto più occupazione? Non avremmo avuto maggiori risposte sotto il profilo delle esigenze di sviluppo dell'impresa? Non avremmo avuto una ricaduta e stime migliori anche sul PIL? Come usiamo i soldi

Proviamo a pensare a questo quando facciamo i nostri provvedimenti d'intervento in materia economica. Proviamo a pensare a come stiamo utilizzando queste risorse. Lasciamo l'egoismo, la propaganda e le tentazioni di prevalere nei confronti dell'avversario politico e poniamoci il problema della risposta che dobbiamo dare al Paese.

come il quadro economico e di finanza pubblica si presenti oggi gravido di incertezze e di rischi. La relazione che oggi discutiamo illustra quindi una fase delicatissima della finanza pubblica, una fase che dovrebbe segnare il passaggio da una situazione strutturale di *deficit* al consolidamento del pareggio di bilancio strutturale. Il risultato del pareggio del risultato del pareggio del 2013 - lo sappiamo bene - è costato moltissima fatica e molti sacrifici agli italiani. È un risultato che oggi, dopo averci portato fuori dalla procedura d'infrazione per *deficit* eccessivo, è di fatto l'unico patrimonio di credibilità che l'Italia può spendere nelle sedi europee, in quelle internazionali e sui mercati. Abbiamo sentito ancora oggi il presidente Letta che riferiva, con la sua immagine dei cattivi dietro la lavagna, come al G20 fossimo usciti da dietro la lavagna. da dietro la lavagna. Ma questo risultato - questo lo dobbiamo sapere bene - non è acquisito per sempre: nei prossimi anni non solo dovremo rispettare il pareggio di bilancio, ma dovremo produrre anche un avanzo primario sufficiente a realizzare quella riduzione del rapporto del rapporto debito/PIL che dovrebbe portarci a dimezzarlo nell'arco di vent'anni. Dunque, gli esami per noi non sono finiti, perché è sulla capacità di onorare questi impegni che saremo misurati e ci sarà dato quel credito che ci è indispensabile se vogliamo destinare le poche risorse disponibili agli investimenti pubblici e non a pagare nuove impennate di tassi di interesse. I dati che abbiamo discusso ieri nel corso dell'esame del disegno di legge di assestamento e la Relazione con cui il Governo dà conto degli effetti prospettici delle misure adottate nei primi mesi di questa legislatura non sono del tutto rassicuranti, come diceva ancora una volta il presidente Azzollini. Innanzitutto, il calo molto sensibile delle entrate fiscali, quasi un punto di PIL, dovuto soprattutto alla diminuzione del gettito IVA, nonostante l'aumento dell'aliquota e, dall'altra parte, un aumento del costo del debito e del livello del debito. Questi dati rischiano di peggiorare ulteriormente, dopo che ieri l'ISTAT ha tagliato ancora le stime relative al PIL per il 2013, portandole a meno 2,1 per cento, anche se molti analisti

Di fronte a questo quadro il messaggio che il peggio è passato e che si può tornare all'andazzo di sempre, cioè a sostenere occupazione e investimenti pubblici nei settori strategici per la competitività (ossia scuola, ricerca, trasformazione digitale e infrastrutture) finanziandoli con spesa pubblica in *deficit* è illusorio e ingannevole. E non solo ciò produrrebbe effetti finanziari nefasti ma, quel che forse è peggio (e su questo dobbiamo riflettere), quel processo di consapevolezza iniziato nella mente e nella coscienza degli italiani con la crisi del novembre 2011 e bloccherebbe sul nascere quel cambiamento culturale il linguaggio della verità con cui il Governo Monti sì è rivolto in quei mesi al Paese ha appena avviato. E non si deve dire che la verità toglie la speranza. Tutt'altro: io credo sia vero il contrario, perché la verità ci può indicare la strada lungo la quale il nostro Paese ha

indispensabili per un nuovo slancio della nostra economia che sia fondato sulla qualità e sulle capacità che il mondo ci riconosce e che non abbiamo perso in questi mesi. Il nostro saper fare artigiano, infatti, la nostra creatività e lo spirito imprenditoriale ancora oggi sono l'unica forza che, grazie alla tenuta delle esportazioni, come dicono i dati macroeconomci, fa reggere la nostra economia. È questo l'orizzonte di speranza con cui l'Italia può afferrare quel vento (che, in verità, a me pare, più che un vento, ancora solo come un piccolo refolo) della ripresa e non disperdere questa nuova opportunità come fece negli anni Duemila, quando, mentre alcuni Paesi europei, in particolare la Germania, grazie alle riforme interne, interne, trasformarono la crescita globale in un robusto e permanente rafforzamento dell'economia interna, l'Italia non riuscì a modificare in nulla il suo *gap* di competitività (motivo per il quale ancora arranchiamo). Il quadro che emerge dalla Relazione presentata dal Governo, che anticipa di poco la presentazione della legge di stabilità, ci dice che non stiamo andando in questa direzione. L'intervento sull'IMU - che avremo modo di analizzare nel dettaglio quando il provvedimento arriverà dalla Camera - è, a nostro avviso, incompatibile con la situazione della finanza pubblica e con le priorità della crescita economica. una misura che va nella direzione opposta a quella unanimemente indicata come essenziale per la crescita, cioè alleggerire il carico fiscale sulle imprese e sui redditi da lavoro oberati da una insostenibile pressione fiscale. i provvedimenti sul pubblico impiego tornano a vecchie logiche di stabilizzazione del precariato, rinviando *sine die* il processo di qualificazione delle amministrazioni pubbliche e il loro graduale ridimensionamento, e tradendo le aspettative di giovani meritevoli che aspettano di avere l'opportunità Ma ciò che più preoccupa, e che la Commissione bilancio sarà chiamata a valutare con estrema attenzione e rigore, sono le coperture finanziarie. Nessuna delle minori entrale e delle maggiori spese correnti decise dal Governo dal suo insediamento viene coperta con riduzioni di spesa. Si spostano tasse da una parte all'altra, si prevedono maggiori entrate IVA quando abbiamo visto la forte riduzione del gettito previsto per l'anno in corso, si aumentano le aliquote delle accise, il cui gettito è anch'esso in forte calo. L'unica misura *pro* crescita è quella dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, processo reso possibile dalla serietà del risanamento finanziario realizzato nel 2012 e dalla chiusura della procedura per *deficit* eccessivo. Il Parlamento si è impegnato su questo tema con un'unanimità di intenti e un'energia che poche volte si sono registrate, e a questa operazione vengono affidate, ora anche dal Governo,

Qui il Governo deve impegnarsi a fondo e si gioca molto della sua capacità di governare e orientare gli apparati burocratici. Infatti, il fallimento, anche solo parziale, di questa operazione determinerebbe conseguenze gravissime in termini economici e finanziari e, soprattutto, minerebbe - io credo irrimediabilmente l'affidabilità dello Stato e il suo rapporto con cittadini e imprese. L'incertezza di molte poste di bilancio e il ritorno all'antico in numerosi interventi segnalano un fatto molto chiaro: non ci sono risorse, e certo stupisce stupisce - questo dobbiamo osservarlo - la velata ramanzina subita dal povero ministro Saccomanni per aver fatto una constatazione tanto vera quanto banale, cioè che, allo stato, per il generoso e anche condivisibile, almeno per alcune parti, accordo Governo-sindacati, i soldi non ci sono. Le risorse possono venire solo dalla crescita, dalla lotta all'evasione fiscale e, come si è detto, dalla *spending review*. Qui però bisogna essere chiari: *spending review* non si può più tradurre con la parola «tagli», ma con la parola con la parola «riforme». Occorre cioè una riorganizzazione di tutte le amministrazioni pubbliche, partendo dalla soppressione di qualcuno dei sette o otto livelli di governo, a cominciare dalle Province che, dopo molti mesi di su e giù, per il momento continuano a stare tutte lì, vive e vegete; occorre spingere sulle liberalizzazioni e sulle privatizzazioni e puntare su incentivi fiscali che orientino i capitali privati su investimenti in infrastrutture, in cultura e, in generale, sui beni di interesse collettivo. Su tutto questo ci aspettiamo una svolta netta e decisa nella legge di stabilità, perché, se è vero che la stabilità politica è un valore, un valore, che rassicura i mercati e rende il nostro Paese più attrattivo, è però altrettanto vero che la stabilità non può essere ottenuta a costo dell'immobilismo. Il voto favorevole che Scelta Civica darà a questa Relazione sta a significare questo:

presentata al Parlamento che sostanzialmente presenta molte carenze e lacune in quello che è l'impatto di rilancio economico del nostro Paese. All'interno di questa Relazione vengono ovviamente evidenziati gli obiettivi e i saldi di finanza pubblica che, se anche parzialmente possono dare un'apparente linea di miglioramento del sistema economico e di quello che è l'andamento del nostro Paese, sicuramente, da parte nostra, non possono essere considerati sufficientemente positivi o comunque avere quella forza di cui il nostro Paese in questo momento ha bisogno per ripresa ha presentato una proposta di risoluzione nella quale porta avanti la richiesta di impegno per il Governo innanzitutto di precisare

che non produce niente e che comunque non può essere oberato da ulteriori imposizioni che affossano quel poco che resta di economia nel nostro Paese. Chiediamo poi di considerare la necessità di potenziare i mezzi e gli strumenti in gestione all'Agenzia del territorio, al fine di incentivare il monitoraggio dei fabbricati catastali, in particolare in certe Regioni dove l'abusivismo è di casa (quindi con un maggior controllo e un monitoraggio del territorio capillare),

Questo è un argomento che ci tocca fortemente, perché è inammissibile che ci siano Comuni che hanno sempre lavorato in maniera corretta, anche tassando maggiormente i cittadini o togliendo loro alcuni servizi pur di arrivare ad una chiusura di bilancio senza*deficit* (o comunque evitando gestioni che non fanno che evidenziare la difficoltà che i Comuni oggettivamente hanno di mantenere certi servizi), e si trovano invece a subire delle tassazioni e delle vessazioni che

signor Sottosegretario, colleghi, le positive notizie che ci ha portato o confermato il presidente del Consiglio Letta dopo l'ultimo G20 certamente danno un ulteriore elemento di lettura per la relazione al Parlamento che oggi ci viene presentata. Ci sono timidi segnali di inversione di tendenza, sia sul fronte della produzione industriale che su quello dell'*export*, ma non possiamo - come abbiamo visto nell'assestamento - non segnalare un crollo dei consumi interni, un calo molto significativo un calo molto significativo del gettito IVA e delle accise dell'energia, che indicano una sofferenza ancora profonda nel Paese. Per cui - lo dico al Sottosegretario credo che più che di ripresa economica imminente sarebbe corretto forse dire che il punto più basso della crisi, iniziata nel 2008, è stato toccato. Riteniamo che, da questo punto di vista, la questione sociale rimanga grave e persistente, e quindi non possiamo che giudicare positivamente il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga per 500 500 milioni di euro anche se mancano - e arriva dalle Regioni con grande forza questo messaggio - rilevanti risorse che dovranno essere trovate entro quest'anno. Altri elementi positivi sono già stati ricordati: l'ulteriore sforzo di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, ad esempio. Di questo condividiamo l'obiettivo di fondo: chiudere questa brutta pagina della finanza pubblica entro il 2014. Un piccolissimo segno nella direzione giusta è arrivato anche sul terreno degli esodati: 6.500 licenziamenti individuali che dovrebbero essere risolti, ma sappiamo tutti che è ancora lunga la strada per arrivare alla soluzione definitiva. Infine, da valutare positivamente è anche il sostegno per l'acquisto della prima casa. prima casa. Non voglio sottrarmi al nodo dell'IMU, che avremo la possibilità di analizzare nel dettaglio quando il provvedimento giungerà al Senato. Credo che qui dobbiamo essere onesti con noi stessi e con il Paese, sottosegretario Baretta. Si poteva fare di più e meglio nella via maestra dell'equità. Non esentare solamente circa 73.000 immobili cosiddetti di lusso è una decisione che contrasta con la crisi in corso e, soprattutto, impedisce di destinare risorse importanti per la crescita e per lenire gli effetti sociali della crisi. Mentre riteniamo che sia stato giusto esentare finalmente i terreni agricoli e gli immobili rurali dall'imposta immobiliare unica. Nel documento presentato dal Governo si rimanda il ridisegno della tassazione immobiliare a successivi provvedimenti. In questa sede vogliamo però cogliere l'occasione per ribadire al Governo alcune nostre indicazioni. Sottosegretario Baretta, lo facciamo senza ricatti, senza proclami, ma con la forza e con la determinazione di una grande forza popolare della sinistra riformista. In primo luogo c'è il tema della riforma del catasto: non possiamo aspettare cinque anni per definire questo problema. In secondo luogo, la *service tax* non può essere un IMU camuffata e quindi dovrà essere individuato un corretto equilibrio tra il corrispettivo per i servizi resi e la componente patrimoniale progressiva degli immobili. Per noi - non ci stancheremo mai di ripeterlo - in questa fase economica chi ha di più deve dare di più. Ultimo, ma non ultimo, l'obiettivo finale deve essere quello di lasciare totalmente ai Comuni i proventi della *service tax* nella prospettiva del «voto, vedo, pago e poi voto di nuovo», valutando l'operato degli amministratori. L'attuale modello fondato sul fondo di solidarietà comunale presenta limiti, rischia di aumentare le tensioni tra i territori e di non risolvere i problemi. Avviandomi alla conclusione, signor Sottosegretario, le rivolgo un invito a controllare bene la previsione di mancato gettito derivante dall'esenzione degli immobili invenduti da parte delle società immobiliari, perché ci pare che quella indicata sui giornali e che abbiamo letto sia largamente sottostimata. Se largamente sottostimata. Se così fosse sono a rischio i bilanci di molti Comuni, soprattutto nelle grandi città. Concludo sottolineando le enormi difficoltà che stanno incontrando Comuni e Province a redigere bilanci di previsione realistici e credibili. Comuni e Province, signor Sottosegretario, che possono essere un formidabile alleato del Governo nella difficile e complessa strategia di ripresa e non devono essere vissuti da parte di alcuni come una sorta di palla al piede. I sindaci e i loro cittadini si attendono segnali di inversione di tendenza nel rapporto tra Stato centrale e autonomie locali, a cominciare, nel documento di stabilità, dall'allentamento del Patto di stabilità per i Comuni. Signor Sottosegretario, da noi continuerà ad avere un sostegno leale. Ci attendiamo, però, maggiore coraggio nella difesa dei principi dell'equità sociale e della coesione territoriale, in una rinnovata alleanza tra Stato ed enti locali virtuosi.

finanze*. Signor Presidente, innanzitutto, per evidenti ragioni di tempo e di approfondimento, rinvio alcune osservazioni di merito sui capitoli relativi all'IMU e alle

Non c'è dubbio che il documento che il Governo ha presentato è la testimonianza della complessità della situazione. Non ce lo neghiamo. Anzi, molto utili ed interessanti sono le osservazioni emerse in questo dibattito. Da un lato, si ha una situazione economica e dei conti pubblici ancora incerta e fragile, suscettibile di rischi non ancora scongiurati. Il peggioramento dell'indebitamento, per le molteplici ragioni che sono state indicate, ne è la prova, ma contemporaneamente sottolineo lo sforzo che stiamo facendo per restare all'interno dei vincoli del 3 per cento che ci hanno consentito di uscire dalla procedura di infrazione. Dall'altro lato, si avvertono tendenze di miglioramento della situazione suscettibili di nuove potenzialità. È esattamente in questa biforcazione fra i rischi ancora presenti di una situazione economica fragile e le potenzialità che si intravedono, sia pure ancora esse stesse fragili, che si inserisce il quadro di scelte di politica economica che il Governo deve fare. Peraltro, è stato citato dagli onorevoli senatori che sono intervenuti e dallo stesso presidente Azzollini che i dati disponibili - da un lato i dati ISTAT di ieri e, dall'altro, i dati di Confindustria di oggi - sono esattamente la testimonianza di questa complessità ed ambivalenza. Non c'è dubbio che nelle scelte che il Governo deve fare dobbiamo focalizzare due aspetti. In primo luogo, lo scorcio del 2013 di fronte al quale - è inutile negarlo - ci sono impegni di finanza pubblica

sulle coperture fosse presente a tutti i colleghi senatori in occasione della discussione che dobbiamo fare sulle scadenze che ci attendono da qui a dicembre. ci sono anche le scelte più approfondite riguardanti il 2014 e oltre che sono inerenti alla legge di stabilità che il 15 ottobre verrà verrà presentata: scelte sulle quali da un lato bisognerà sicuramente avere attenzione alla finanza locale. Prima la collega senatrice della Lega lo ha ricordato: un'attenzione particolare agli sforzi che gli enti locali hanno fatto in questi anni

Dall'altro lato, sicuramente quella piattaforma che le parti sociali hanno presentato, pur nella complessità che essa manifesta, va presa in considerazione. Con questi due elementi noi dobbiamo costruire una legge di stabilità ‑ la senatrice Lanzillotta ha chiaramente ragionato su alcune di queste cose ‑ che deve imprimere quell'elemento di svolta verso la ripresa. Da questo punto di vista (ed è la seconda e ultima considerazione che voglio fare) non c'è dubbio che il perno di questa prima fase è stato quello dei pagamenti della pubblica amministrazione. Se ne vedono gli effetti. Se ci sono ritardi, noi siamo in una collegialità di Governo per affrontarli; ma non c'è dubbio che aver deciso uno stanziamento di 40 7 (tendenti a 10), e per quest'anno 27,2, è un segnale molto concreto, che è già in atto. Si può discutere dei ritardi, ma si deve percepire che questa dinamica è già in movimento e sta scendendo rapidamente dal centro alla periferia. a porre la questione di approfondire meglio il rapporto che ci dovrà essere tra questa entità importante di gestione della finanza pubblica e gli obiettivi strategici che ci attendono, Non c'è dubbio che, come già si vede, la manovra pone, da un lato, emissione, ma dall'altro anche nuove possibilità di entrate che, se adesso abbiamo coperto per far fronte ad esigenze immediate, in prospettiva possono costituire un ristoro della stessa finanza pubblica. non risolutivo può intravvedersi un primo accenno di riflessione e di risposta alla questione cui lei, presidente Azzollini, ha accennato. In conclusione, signor Presidente, devo dire che però una risposta compiuta a tutte queste problematiche arriverà tra pochi giorni, quando, entro il 20 di questo mese, verrà consegnata la Nota di aggiornamento sul Documento di economia e finanza, che, come loro sanno, è il presupposto per una discussione sulle scelte di merito che faremo nella legge di stabilità. Con questo spirito, e avendo ascoltato il dibattito, il Governo esprime un parere favorevole sulla proposta

Poiché il Governo ha dichiarato di accettare la proposta di risoluzione n. 3, decorre da questo momento il termine di trenta minuti per la presentazione di eventuali emendamenti ad essa riferiti. Le dichiarazioni di voto avranno luogo nella Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri in quest'Aula, proprio come adesso, intervenivo per denunciare un fatto gravissimo: la morte di una giovane dottoressa. Stasera intervengo invece perché nonostante la drammaticità la drammaticità di un incidente stradale che ha visto protagonisti due findanzatini nel comune di Cazzano Sant'Andrea, alcune sere fa le cose sono andate in modo diverso, fortunatamente in modo diverso. Forse l'alta velocità, forse la perdita di controllo dell'auto, sta di fatto, signor Presidente, che il mezzo meccanico esce di strada, sbatte violentemente contro un muro in cemento armato e l'auto comincia a prendere fuoco. Quando l'auto ribaltata era già in fiamme, giungono sul luogo dell'incidente Jacopo, 18 anni, e subito dopo Nicola, di 20. Le loro strade si sono incrociate probabilmente per un disegno divino. disegno divino. L'istinto, la voglia di salvare ragazzi come loro: hanno trascinato fuori dall'abitacolo prima Stefania e poi Giordano, privi di sensi ed impossibilitati a salvarsi da soli. Celermente sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e le autoambulanze; si sono recati sul luogo dell'incidente, ma l'auto era completamente carbonizzata.

avranno per sempre la mia riconoscenza, senza di loro e il loro intervento ora avremmo due funerali. Chiudendo, signor Presidente, colleghi, siamo abituati a sentir bistrattare i ragazzi; li chiamiamo schizzinosi, svogliati, bamboccioni, indifferenti. Una mite serata di fine estate, interrotta da un terribile botto, ha messo invece in luce i bravi ragazzi, quelli che non ci aspettiamo e che non hanno l'onore della cronaca. oscurati da luoghi comuni, troppi luoghi comuni. Questi ragazzi hanno messo a repentaglio la propria vita per salvare quella di due ragazzi come loro. Hanno fatto quello che ognuno di noi dovrebbe fare e troppe volte non viene fatto. I genitori, la nostra comunità e il mio Gruppo parlamentare vi sono grati per il coraggio che avete messo a disposizione di due ragazzi come voi e questo rincuora tutti: un gesto di assoluto altruismo che rincuora tutti di fronte a tanto egoismo e indifferenza che che contraddistinguono la società di oggi. Gesti come il vostro infondono una nuova speranza per una società migliore. Grazie Jacopo, grazie Nicola e auguri ai due ragazzi, nella speranza che guariscano presto. Essi saranno presto ospiti del Senato

«Gentile senatrice Sara, chissà mai se leggerà in Senato quello che penso e scrivo io, ma pure qualche milionata di italiani. Mi tratterrò dal dire parolacce, che poi le fanno problemi! Ho visto ieri che di nuovo avete beccato una senatrice che votava per uno che non c'era... n'altra volta... ma quanti ce ne stanno di sti pianisti? E pure era la terza volta che la beccavate a fa sta zozzeria de votare per un altro... ma dopo tre volte non dovrebbe scattare il cartellino rosso e l'espulsione? Ma che punizione gli danno? A me mi sembra che chi vota per uno che non c'è, quello che non c'è non perde i soldi della giornata, o giù di lì. Come se fosse al lavoro... allora gli dica che se io timbro il cartellino del mio collega all'orologio della mia fabbrica a me mi fanno un mazzo così, mi sospendono dal lavoro e mi fanno una multa tanta. E vogliono pure cambiare la Costituzione, questi senatoroni qua! E poi... che so, quel giorno che uno manca l'accusano che fa 'na festina a base di coca in hotel insieme a due signorine allegre e una tra un po' ce rimette le penne... lui po' dire che non era lui, perché era in Aula a votare... e ha le prove del suo voto... E se magari un senatore... diciamo che lo accusano che quel giorno ha dato una mazzetta de 5 mijoni di euro per corrompere un collega che gli fa un favore... ebbene, lui può dire che noooo, perché stava a votare. Non si può fare, è ora de farla finita, chi vota per un altro va allontanato e multato alla grande!!! Ci sono stati seduti su quelle poltrone gente come De Gasperi, la Iotti, Moro e Tina Anselmi. *(Applausi dal Gruppo M5S).*Anche qualcuno con idee diverse dalle mie,

Meno male che voi li mettete sulla rete a sti furboni. Senatrì, visto che tanto non gli fanno niente a sti Mozart, fa' una cosa bella, mettiti vicino una scarpa bella grossa, del 44 che è il mio numero di piede, e la prossima volta tiraje na' scarpata... se non fanno niente a loro, non vi faranno niente manco a voi, che tutto sommato fate una cosa che v'ha chiesto un cittadino onorevolissimo per davvero. E mi dico... ma se ci fosse ancora Pertini... oooh se ce fosse Pertini... la scarpata gliela tirerebbe lui!!»

desidero porre all'attenzione dell'Assemblea due episodi apparentemente lontani tra di loro, ma che hanno un punto in comune: la violenza sulle donne. Il primo è l'uccisione a coltellate di una collega medico, la dottoressa Paola Labriola, Non posso che esserne addolorato, sia come persona che come collega. In questo caso si tratta dell'ennesima violenza contro una donna da parte di un attentatore con una coscienza alterata. Ciò può accadere a chiunque, ma una donna è più esposta, in quanto al suo aggressore può sembrare una preda più facile. Dobbiamo però soffermarci sul fatto che in psichiatria la violenza è molto rara, se confrontata con gli atti violenti della cosiddetta gente normale: non cadiamo quindi nella banalizzazione, che stimola molte fantasie popolari, alla ricerca di capri espiatori per superare il peso di un mondo sociale sempre più ostile. Ricordiamo invece che la violenza improvvisa è difficilmente gestibile, ma anche che basterebbe la presenza di un collega per scoraggiare il malintenzionato. Oggi questa semplice precauzione è difficile da mettere in pratica, a causa dello stato di abbandono in cui versano il Sistema sanitario nazionale e, in particolare, i dipartimenti di sanità mentale. Risolvere il problema non vuol dire mettere in atto misure di ordine pubblico, ma dare attuazione a politiche sanitarie giuste e utili. Quindi, questa morte va inserita nell'ambito della responsabilità politica e morale di chi ha permesso che sistemi di cura così delicati, come quelli relativi alla salute mentale e alle dipendenze, fossero sempre più indeboliti da restrizioni di mezzi, di organico e finanziarie. È dunque indispensabile in questo momento sbloccare il blocco del *turnover* che ha paralizzato questi servizi. Un secondo esempio di violenza sulla donna è quello perpetrato in questi giorni: mi riferisco alla notizia che una nostra collega deputata non ha potuto usufruire di un servizio dovuto per legge, quale la prescrizione della cosiddetta pillola del giorno dopo, presso l'ambulatorio di Montecitorio. Questo per il semplice motivo che il medico ha risposto di no per motivi di coscienza e anche il medico del turno successivo era obiettore di coscienza, come tutti gli altri: si tratta di colleghi medici che lavorano alla Camera dei deputati. Ricordiamo che l'11 giugno 2013 la Camera dei deputati ha approvato sette mozioni, presentate dai diversi Gruppi parlamentari, in cui si invitava il Governo a dare piena applicazione alla legge n. Io stesso ho presentato un disegno di legge, che spero venga appoggiato dai vari Gruppi parlamentari, per fare in modo che questo servizio sia assicurato in ogni ospedale pubblico e in ogni struttura privata accreditata. Non è pensabile che ciò non sia garantito perché tutti i medici del servizio sono obiettori: se l'obiezione è un diritto, di esso non si può abusare, soprattutto se lo si fa per motivi di carriera interna, più che per convinzione religiosa o ideologica. La legge n. 194 è sempre più osteggiata, a tutto danno dei diritti delle donne.